Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge: *dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Ministri degli affari esteri, della difesa, dell'interno, della giustizia

di fare di ogni decreto una sorta di decreto *omnibus* e comunque di introdurre argomenti di grande rilevanza politica nella navetta dei decreti-legge presentati dal Governo.

provvedere. Mi sembra conseguente a questa pratica che di fatto si sta seguendo in entrambe le Aule del

emendamento

Senatore Perduca, lei ha sollevato un'obiezione che è condivisa da tutta l'Assemblea. Mi dicono che c'è un problema e che stanno lavorando per cercare di risolverlo.

come è noto, impone che gli abbonati inseriti negli elenchi stessi possano essere utilizzati come potenziali consumatori solo ed esclusivamente per certe finalità.

fare una semplice osservazione. Fermo restando quanto stabilito in sede giurisdizionale in merito a questo argomento (mi riferisco alla Corte costituzionale e al TAR), ritiro l'emendamento 20.4, anche sulla base delle affermazioni incontrovertibili che, in modo assolutamente rassicurante, ha reso il Governo per il tramite del ministro Ronchi, con l'impegno di disciplinare questa materia riconducendola ad un ambito di assoluta regolarità e conformità alle disposizioni vigenti. D'accordo con gli altri colleghi firmatari, i senatori Cursi e Battaglia, chiedo che venga accettata - è questa la valutazione che pongo al relatore e al Governo la trasformazione dell'emendamento 20.4 in un ordine del giorno nel quale si rinnovi l'impegno che lo stesso ministro Ronchi in sede di replica ha rilasciato all'Assemblea con la piena disponibilità a procedere alla revisione della normativa in tempi assolutamente certi. Ove questa richiesta dovesse essere

per comunicazioni di mercato. Esiste una normativa, sotto la tutela dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, che impedisce l'utilizzo dei tabulati salvo esplicito consenso;

Questo rinvio di ulteriori sei mesi, rispetto ad un rinvio che già vi fu in un altro provvedimento, proroga una situazione selvaggia come quella attuale e non mette fine ad un regime assolutamente contrario a quella tutela della *privacy* cui tutte le nostre norme ormai si ispirano. Il testo

per gravare, di fatto, sugli abbonamenti dei cittadini; non solo, dacché questo registro, che disporrà di un potere di mercato enorme, non sarà controllato, se non

è regolata dalla direttiva 2002/58/CE che, all'articolo 129, stabilisce che i dati personali degli abbonati inseriti negli elenchi telefonici possono essere utilizzati per finalità di mera ricerca dell'abbonato per comunicazioni interpersonali. Ora, già

20.0.502. In considerazione della politica comunitaria, volta a ridurre al minimo le conseguenze negative della produzione e della gestione dei rifiuti per la salute umana e l'ambiente, risulta di primaria importanza chiarire la distinzione tra ciò che è rifiuto e ciò che non lo è, il e ciò che non lo è, il tutto al fine di ridurre l'uso generalizzato di risorse e promuovere l'applicazione pratica della gerarchia dei rifiuti. La strategia comunitaria definisce come priorità principale della gestione dei rifiuti la prevenzione ed il riutilizzo dei materiali, per introdurre un approccio che tenga conto dell'intero ciclo di vita dei prodotti, al fine di preservare le risorse naturali, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle stesse e migliorandone l'efficacia dello sfruttamento attraverso il loro completo utilizzo. Per il perseguimento di tali obiettivi, al fine di dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea hanno adottato la direttiva

Ritenendo che il solerte recepimento di tale direttiva da parte dell'Italia possa assicurare il chiarimento di alcuni contesti normativi, al momento di difficile interpretazione, oltre che favorire l'utilizzo di materiali ad oggi destinati a discarica, con un conseguente impatto concreto sul settore produttivo ed economico, si considera fondamentale perseguire tale obiettivo con energica celerità. In particolare, risulta di primaria importanza chiarire quando Grazie, Adeguare la legislazione italiana al concetto di sottoprodotto come definito dalla direttiva comunitaria permetterebbe, da un lato, di eludere la confusione tra i vari aspetti della definizione di rifiuti e, dall'altro, di valorizzare materiali in possesso di caratteristiche idonee per l'utilizzo nei normali cicli produttivi ed industriali, (anche di altre attività) attualmente trattati come rifiuti. Un esempio concreto è dato dai residui della lavorazione lapidea a fini ornamentali che, nella maggioranza dei casi, mantengono inalterate le caratteristiche del materiale originario anche al termine del processo produttivo e potrebbero pertanto essere impiegati in sostituzione dei materiali di cava di sabbia e ghiaia nella produzione di aggregati per l'edilizia. Per queste ragioni, signor Presidente, chiedo l'approvazione dell'emendamento 20.0.502 che

garbata veemenza dai senatori dell'opposizione. Vorrei sottolineare che una gran parte delle telefonate indesiderate che si ricevono oggi dipendono dal dal difettoso funzionamento delle norme oggi in vigore, a parte la proroga stabilita nell'ambito del decreto "milleproroghe". "milleproroghe". Quando queste norme saranno pienamente in vigore (parliamo della fine di maggio, non di una data lontana), coloro che non vorranno ricevere telefonate indesiderate di promozione commerciale, di vendita e così via in un registro, con una telefonata o con un messaggio di posta elettronica. Una volta che saranno iscritti a questo registro, non potranno essere chiamati per ragioni commerciali. Oggi, in teoria, c'è una norma più garantista, in pratica, questa norma non è efficace, perché molti hanno dato l'assenso a ricevere queste chiamate, o

Pertanto, la situazione di oggi è molto simile a quella che viene preconizzata, a mio avviso in modo non coerente con ciò che tale emendamento propone, per il futuro. L'emendamento 20.0.500 prevede altresì cui viene individuato il soggetto presso il quale viene collocato tale registro, e su di esso vigilerà il Garante per la riservatezza dei dati personali: questo è l'aspetto essenziale che garantisce la riservatezza. Ricordo altresì che si tratta di un sistema in vigore in molti Paesi, in particolare negli Stati Uniti e in Gran Bretagna, dove la promozione telefonica

Prego l'obbligo di segnalazione è previsto nel caso in cui vi siano ulteriori reati, e quindi è già previsto dall'ordinamento. Nel caso in cui invece si tratti di risorse scudate, si tratta di un comportamento lecito, quindi l'obbligo diventa superfluo. Sotto questo profilo,

si chiede di acquisire il parere del Garante anche in ordine al regolamento che disciplina l'istituzione del registro per le opposizioni al trattamento dei dati. Questa è una precisazione che riteniamo estremamente importante, perché questo è un ruolo affidato al Garante dalla normativa comunitaria: comunitaria: è una attribuzione in relazione alla tutela di un diritto fondamentale quale quello alla protezione dei dati personali. Ricordo solo incidentalmente che la Carta di Nizza, all'articolo 8,

conferendo loro un ruolo di assoluta rilevanza nella tutela di tale diritto. Ora, anche nell'ottica della norma che viene proposta dalla maggioranza e dal Governo, è incomprensibile questo rifiuto di richiedere, per tali situazioni, il parere del Garante

Grazie,

da 20.000 a 10.000 euro. Però, al contempo, proprio per l'introduzione del nuovo regime, molto più rigido (per cui possono essere contattati soltanto quelli che non hanno espresso il proprio diniego) e proprio perché la violazione è più grave,

la votazione).* Prego il senatore Azzollini di essere più calmo con la sua mano sinistra.

Signor Presidente, colleghi, mi rendo conto che siamo a conclusione di una giornata di lavori particolarmente estenuante. Abbiamo votato alcune centinaia di volte su argomenti, collega Incostante, molto diversificati l'uno dall'altro. Abbiamo parlato delle questioni più incredibili. Vi chiedo un momento di attenzione, e lo chiedo in particolare al relatore ed al Governo.

sussulto. Questa è una di quelle norme che incidono sulla qualità della vita dei cittadini del nostro Paese, direttamente e indirettamente. Non so se è chiaro, colleghi, di che cosa esattamente si tratta. tratta. Ognuno di noi, anche per sua esperienza personale, sa che ormai nel nostro Paese è estremamente diffusa una prassi per la quale alle ore più incredibili del giorno, e qualche volta anche della sera,

queste incredibili strutture che si chiamano *call center* e che guadagnano, spesso in condizioni di grande precarietà, uno stipendio da fame per fare telefonate che sono francamente molto gravi.

passare da un sistema nel quale è richiesto l'esplicito consenso per ricevere delle telefonate, come quello teoricamente in vigore oggi nel nostro Paese,

il passaggio ad un sistema che presume il consenso dei clienti avrà sicuramente una gravissima incidenza sulla serenità della vita delle nostre comunità. Trovo francamente incredibile

occorre riflettere, vi chiedo di votare serenamente contro l'emendamento del relatore. Avremo tempo e modo per affrontare in modo congruo una riforma così importante per il nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo

mi permetto di dire al senatore Bianco, nei cui confronti ricambio la stima, che una cosa è il sistema di *opt-in* e *opt-out* per il trapianto di organi, ben altra cosa, invece,

manifesterà solo disappunto, alla seconda si arrabbierà, alla terza o alla quarta si ricorderà, perché la cosa verrà resa pubblica, che esiste la possibilità di iscriversi ad un registro

di molti di noi -, senza che ne siano a conoscenza, è proprietà di qualcuno, lo ripeto, che ha acquisito a suo tempo il diritto a chiamarli sulla base del silenzio assenso, per cui non possiamo certamente descrivere la situazione odierna come ideale

va a finire che il senatore Malan adesso vorrebbe convincere l'Assemblea che questo emendamento molesto

che voi non avete voluto in questo Paese, svuotando l'azione di classe di contenuto, rinviandola alle calende greche e sostituendola

e anche del codice del consumo. Lei, senatore Malan, lo ha ritirato in Commissione e ha fatto il *blitz* nell'Aula affinché le associazioni dei consumatori e gli stessi

dunque, conquistarsi la propria pace lottando contro le macchine perché, tra l'altro, lei istituisce anche il diritto alle molestie tramite *fax*. Forse non se ne é reso conto: si può molestare anche tramite *fax*. Ancora una volta, in deroga alla disciplina del codice della *privacy*,

Si tratta, infatti, della riproduzione letterale di un'importante parte della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti che ha favorevolmente sorpreso tutti i Paesi membri e soprattutto tutte le forze politiche presenti in questo Parlamento attraverso giudizi espressi in Commissione ambiente. La direttiva innova profondamente nell'identificazione della qualifica del sottoprodotto, oltre ad avere tanti altri pregi nel suo contenuto generale. La Commissione ambiente e poi il Senato l'hanno immediatamente indicata nell'ambito della legge comunitaria 2008 come una direttiva da recepire con assoluta urgenza.

definizione è attesa da tutto il mondo produttivo nazionale e, soprattutto, dagli artigiani e dalle medie, piccole e piccolissime imprese che hanno sempre avuto delle difficoltà

ha indicato come una delle direttive da recepire con immediatezza nell'interesse della collettività nazionale.

entro giugno del prossimo anno il Ministero dell'ambiente dovrà predisporre i decreti legislativi che dovranno affrontare anche i temi della qualificazione di ciò che è sottoprodotto e di ciò che, invece, va considerato rifiuto. si sa - quelli che apparirebbero sottoprodotti (penso ai materiali inerti, ma contaminati) sono stati utilizzati anche per costruire delle scuole (mi riferisco al caso recente di Crotone), penso che di tutto ci sia bisogno tranne che di affrontare questo tema delicato con leggerezza ed approssimazione.

delle operazioni finanziarie relative al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo sarebbe in vigore. Ricordo che la norma introdotta con lo scudo fiscale ha inserito la deroga all'obbligo di segnalazione. Per quale motivo introducete la deroga all'obbligo di segnalazione per operazioni sospette relative al terrorismo e alla criminalità organizzata? Cosa c'entra con lo scudo fiscale? Per quale motivo lei ha dovuto dare una giustificazione che è offensiva per il Parlamento, e lei lo sa benissimo? Dite chiaramente che volete aiutare la mafia e il terrorismo!

prevedeva l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette per riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Con lo scudo fiscale avete introdotto la deroga all'obbligo di segnalazione per le operazioni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo. Noi chiediamo di reintrodurre questo obbligo, in linea con la direttiva europea, in un decreto‑legge recante disposizioni per l'attuazione di obblighi comunitari. Voi rifiutate un emendamento che è in linea con gli obblighi comunitari, favorendo mafia e terrorismo. Non dica menzogne!

l'accumulazione di capitale derivante da attività criminose di stampo mafioso, ovvero depositi finanziari che siano collegati all'esercizio di attività terroristiche. Penso che un emendamento di questo genere, accolto dal Governo e dal relatore, sia non solo perfettamente coerente con la natura e l'oggetto di questo decreto, ma sia anche

invito il senatore Fluttero a ritirare l'emendamento, per poterlo presentare, con più forza, con riferimento

e parere favorevole Presidente, il Gruppo dell'Italia dei Valori esprimerà voto contrario sull'emendamento

interpretazioni che possano ingenerare confusione. Avevamo apposto la nostra firma Grazie,

un principio generale come quello che questa disposizione introduce nel nostro ordinamento, ossia la liberalizzazione e sostanziale privatizzazione della gestione dell'acqua in assenza di un sistema di garanzia indipendente e adeguato.

quanto meno discutibile. Paghiamo ancora la privatizzazione delle autostrade con aumenti di tariffe assolutamente sproporzionati ed assenza totale di investimenti. In tempi recenti, come tutti ricordiamo, abbiamo registrato abusi della concessione della rete telefonica privatizzata.

senza la minima riflessione da parte del Parlamento ed utilizzando i nostri Regolamenti, quindi escludendo dalla discussione un emendamento che prevedeva l'istituzione di un'autorità di garanzia.

Tutti noi siamo favorevoli alla liberalizzazioni, e lo siamo quando servono anche alle privatizzazioni, ma in un mercato regolato: privatizzare l'acqua in un mercato non regolato, signor Presidente, è una cosa gravissima che nessuna democrazia moderna

Presidente, apprezzo gli sforzi effettuati per ricondurre a ragionevolezza una tematica così importante.

pubblico e non privato.

invece un tema di primaria importanza. Lo dicevo questa mattina e non voglio ripetere quanto ho detto. È ovvio che, di fronte a una questione come questa, chi si interroga seriamente su questa partita può scegliere strade diverse. È la strada che hanno scelto con piena onorabilità e anche con la necessità che ad essi si porti il massimo del rispetto

- come si suol dire, che passi una proposta, quella del Governo, che, di fatto, lascia insolute le grandi questioni democratiche che attengono al tema della gestione e della proprietà della risorsa idrica,

che la proprietà non può che essere pienamente pubblica, che la gestione delle risorse sia autonoma in quanto all'organizzazione della società privata, ma che l'accesso universale, i prezzi, la qualità della fornitura e la stessa accessibilità siano garantiti dal pubblico e corrispondano a diritti di cui le istituzioni pubbliche competenti hanno la responsabilità. Credo che noi abbiamo apportato un miglioramento al testo del Governo e che, in qualche modo,

di una migliore soluzione di questa questione che, altrimenti, sarebbe stata approvata dalla maggioranza, vista la capacità di ascolto dimostrata normalmente nei confronti di questo tema, in piena autonomia e - aggiungo - con disprezzo e pericolo pericolo per le ragioni che abbiamo ritenuto avessero invece la necessità di trovare nella legge, in questa legge, una piena e chiara affermazione. Presidente, colleghi senatori, il provvedimento che stiamo discutendo contiene indubbiamente una norma di portata storica perché la riforma della gestione dei servizi pubblici locali ed una loro maggiore liberalizzazione è tema che da anni veniva discusso in Parlamento, in varie legislature, con diverse maggioranze e diversi Governi, senza trovare una soluzione. Il tema è, ripeto, molto complesso: si tratta di garantire meno sprechi, una gestione più efficiente ed anche attenta al mercato, di evitare monopoli locali o monopoli di estensione crescente sul territorio, ma anche di garantire ai cittadini quei servizi a condizioni economiche accettabili, soprattutto per beni indispensabili - stiamo parlando dell'acqua La nostra intenzione nel votare a favore di questo provvedimento (che contiene molti elementi, ma che adegua anche ad esigenze europee i servizi pubblici locali) è quella di una svolta di modernità che garantisce una serie di diritti.

che abbiamo dovuto dare ascolto ad alcune sollecitazioni. Riteniamo che l'impianto del provvedimento sia assolutamente valido, ma che questo emendamento, presentato dal senatore Bubbico, confrontatosi rappresentate in Parlamento (e da questo nasce il nostro voto favorevole), scandisce in maniera ancor più chiara che l'apertura a diverse forme di gestione non mette in discussione la proprietà pubblica del bene acqua e la necessità che esso venga erogato nel territorio Grazie, dal suo punto di vista e con le sue valutazioni, che come maggioranza si debba rivendicare la capacità dell'ascolto. È stata posta una questione nel Parlamento e fuori: esistono associazioni, movimenti, *e-mail* che arrivano a tutti noi e che invitano ad un'attenta riflessione su questo tema delicato. che l'emendamento Bubbico renda ancora più chiara questa materia. Quindi abbiamo dichiarato - e lo ribadisco anche ora - il nostro voto a favore. Credo che trovare dei segmenti di condivisione di percorso su temi di interesse generale sia una scelta saggia a favore della quale noi voteremo con grande convinzione.

credo che quella sia la sede più opportuna e giusta al fine di poter prevedere, con un ragionamento profondo e condiviso, questo argomento. Presidente, voglio anzitutto ringraziare i colleghi, il relatore ed il Governo per l'attenzione che questo mio emendamento ha suscitato.

di riciclaggio o terrorismo, deve essere segnalata. Questa norma, indiscutibilmente, resta, ma la dizione precedente potrebbe far sorgere l'opinione errata che si debbano segnalare tutte le operazioni che vengono effettuate.

Ma è esattamente questo il punto! Lo scudo fiscale può essere uno strumento attraverso il quale si attuano proprio quelle operazioni che sono soggette a registrazione, quindi se non ci intendiamo su questo punto è ovvio che non ci intendiamo neanche sull'emendamento. L'intenzione dell'emendamento del senatore Li Gotti era esattamente questa: fare in modo che lo scudo fiscale non possa essere in nessun modo un

carico agli intermediari finanziari l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette relative al riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Lo scudo fiscale ha introdotto la deroga a questo obbligo di segnalazione.

anche nei casi di applicazione dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2009, cioè anche nei casi di applicazione dello scudo fiscale, rimanga fermo l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

Presidente, colleghi, il decreto-legge che abbiamo esaminato insieme a disposizioni che assicurano l'adempimento di obblighi derivanti dalle norme comunitarie e dall'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia ovvero da procedure d'infrazione pendenti, contiene in verità diversi interventi - troppi - volti a risolvere controversie che sussistono ormai da molti anni e per le quali si sarebbe potuto intervenire con un normale disegno di legge. legge. Si dovrebbe, quindi, chiarire se il fondamento della decretazione di urgenza possa consistere semplicemente nella circostanza che sono scaduti i termini per adempiere. Sarebbe più opportuno che il Parlamento esaminasse in tempo utile il disegno di legge comunitaria annuale, secondo quanto indicato anche da un ordine del giorno approvato dal Senato.

e al fine di consentire alla 14a Commissione di operare l'esame di tutta la materia di matrice comunitaria. Nella realtà, il provvedimento in esame evidenza una profonda disattenzione dell'Esecutivo verso le politiche europee complessivamente. Esso contiene alcune previsioni che hanno poco a che fare con l'esigenza di porre rimedio a condanne che concludono procedure d'infrazione. L'articolo 15, del quale abbiamo tanto opportunamente, ma invano discusso, reca norme che intervengono in modo che non esito a definire grossolano sulla materia delicata dei servizi pubblici locali, ponendo in questione l'equilibrio su cui si fonda il funzionamento di molte società miste che gestiscono tali servizi. I servizi pubblici locali rappresentano un settore strategico per la modernizzazione del Paese: riteniamo che la riforma presentata dal Governo sia insufficiente a rispondere ai problemi di questo settore. Abbiamo presentato un emendamento che era interamente sostitutivo dell'articolo 15 proprio perché il provvedimento del Governo è un semplice aggiustamento normativo e non una risposta esaustiva al problema. Il monopolio che continuerà ad esistere dopo l'approvazione dell'articolo 15 avrà soltanto un risultato: gli utenti finali, cioè i cittadini, pagheranno sempre di più i servizi pubblici fondamentali. Questa riforma improvvisata, frutto di un compromesso al ribasso tra i partiti della maggioranza, affossa ancora di più il settore dei servizi pubblici. I servizi pubblici locali costituiscono una leva formidabile per soddisfare i bisogni delle famiglie e per venire incontro alle sollecitazioni provenienti dal mondo delle imprese. «Servizi migliori a prezzi più bassi» non dovrebbe essere soltanto una formula vuota da agitare a fini propagandistici, ma un vero obiettivo da perseguire in tutta la sua concretezza. Per fare questo però occorrerebbe muoversi in due direzioni: in primo luogo bisognerebbe prevedere che l'affidamento del servizio avvenga in via ordinaria tramite gara pubblica; in secondo luogo è necessario affrontare il vero nocciolo della questione ovvero il conflitto di interessi tra ente regolatore e soggetto gestore, che contraddistingue gran parte degli affidamenti esistenti, incentivando gli enti locali affinché escano finalmente dal mercato dei servizi pubblici locali. In una parola, occorre convincersi della necessità di aprire al mercato e soprattutto alla concorrenza l'intero settore. Di tutto questo, però, nelle proposte del Governo non c'è assolutamente traccia. Si continua a prediligere la via più breve della normativa di principio senza preoccuparsi di comporre una trama dal senso veramente compiuto, essenziale per gli operatori, attraverso la predisposizione di forme di integrazione con la disciplina settoriale. Si salvano senza tentennamenti gli affidamenti diretti a società *in house*, limitandosi a prevedere un inutile obbligo di motivazione a carico dell'ente locale; inutile perché non è accompagnato da strumenti, anche sanzionatori, volti a verificare l'effettiva sussistenza delle ragioni che ostano all'utile ricorso al mercato. neanche pensare che basti l'invio della relazione all'Autorità garante della concorrenza del mercato o alle Autorità di settore, ove costituite, per il rilascio di un parere successivo alla scelta e, comunque, non vincolante. Si fa soltanto finta di credere nel principio della proprietà pubblica delle reti. Che si tratti di una finzione, infatti, è oltremodo palese nella volontà di non definire concrete modalità anche finanziarie per addivenire a questo risultato. È evidente che lo sviluppo economico, civile e sociale delle collettività territoriali è promosso soprattutto attraverso la disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica; una disciplina che cade in un momento particolare della vita sociale ed economica dei diversi territori. Essi, infatti, tra non molto dovranno confrontarsi con il federalismo fiscale e con il problema di garantire il diritto di tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi pubblici locali nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere *e*) a meno che non si sia costretti a ipotizzare una sorta di gabbie fiscali, rapportando così il fisco alla quantità e qualità dei servizi a disposizione degli utenti e sancendo con ciò stesso una evidente disparità di diritti fra cittadini di diversi territori, disparità inconciliabile, naturalmente, con il dettato dell'articolo 3 della nostra Costituzione, ancora vigente, mi pare. Inoltre, si affronta soltanto di sfuggita e con una certa improvvisazione il problema del regime delle società quotate; si persevera diabolicamente sulla strada di concepire i servizi pubblici locali in chiave eminentemente localistica. Non serve essere particolari conoscitori delle realtà delle amministrazioni locali e regionali per rendersi conto del fatto che la possibilità per le Regioni e gli enti locali di ridefinire i bacini di gara per i diversi servizi non è altro che l'ennesimo *spot* e come tale resterà lettera morta. Per queste semplici ma risolutive ragioni, il Governo avrebbe dovuto far propria la proposta di stralcio avanzata non soltanto dal nostro Gruppo, ma anche dalle altre forze di opposizione, nonché da vasti settori del mondo economico e delle associazioni dei consumatori. La riforma dei servizi pubblici locali è un tassello fondamentale per restituire competitività al Paese, per contribuire al rilancio del nostro sistema produttivo e per risollevare il potere d'acquisto delle famiglie. Pensare di farlo attraverso una normativa indubbiamente improvvisata è il modo migliore per affossare definitivamente qualsiasi proposito realmente riformatore dell'intero settore e per frustrare ancora una volta le aspettative delle imprese e delle famiglie, soprattutto in quelle Regioni del Sud Italia (ma non solo) ancor meno dotate di servizi e di infrastrutture. Dobbiamo rilevare anche la scarsa sensibilità del Governo sulla salvaguardia delle competenze delle Regioni e delle Province autonome.

impropriamente in questo decreto-legge, potrebbe avere, per esempio, sulla complicatissima vicenda dell'acquedotto pugliese. L'inserimento, con emendamenti del Governo, di provvedimenti di grande rilievo estranei alla materia specifica del decreto-legge, l'attenzione ancora una volta sbilanciata verso l'agricoltura di una sola parte del territorio nazionale sono tutti motivi che inducono tutto il nostro Gruppo a esprimere un voto convintamente contrario.

che siamo stati costretti a votare. Sono costretto però ad attirare l'attenzione dell'Aula su un tema che dovrebbe diventare argomento di riflessione e cioè la falsa bicameralità del nostro lavoro. le Camere hanno 60 giorni per convertire in legge il decreto, che pertanto scade il 24 novembre.

pur potendo contare su circa cinque settimane di lavoro, l'esame effettivo dei testi è stato concentrato in pochissime caotiche ore.

è poi approfittato della situazione per allargare lo scudo fiscale al punto da introdurre nel decreto l'espressa disapplicazione delle convenzioni internazionali sul riciclaggio e l'antiterrorismo.

della privatizzazione di un bene comune fondamentale. Trascuro altre questioni, anche perché vi sono già stati specifici, validissimi interventi, sul quadro della disorganicità interna di questa falsa riforma del servizio pubblico, ma sulla questione dell'acqua è impossibile chiudere gli occhi. Noi abbiamo di fronte una situazione drammatica. Come è dimostrato da una vastissima pubblicistica mondiale, l'acqua è già diventata un fondamentale motivo di guerra.

francesi e tedeschi che illustrano tutti una pericolosità crescente del tema acqua dal punto di vista del rapporto tra i popoli, tra ricchi e poveri e tra Nord e Sud del mondo. L'elemento è dirompente, voi lo volete affrontare imponendo in modo sgangherato un processo opaco di privatizzazione sotto la logica ipocrita secondo cui l'acqua resta pubblica ma la gestione diventa privata.

fatto che la privatizzazione fa decuplicare i prezzi dell'acqua, li fa moltiplicare, peggiorando la qualità dell'acqua e senza dare alcuna garanzia sul controllo delle reti degli acquedotti. C'è un processo di progressivo, inarrestabile peggioramento della della captazione, della diffusione e della distribuzione di una risorsa comune fondamentale e tutto ciò in nome di una privatizzazione che consegna ad un pugno di soggetti incontrollabili, una nuova specie di roditori privati che si apprestano a divorarla, una fondamentale

il caso di Roma. Voci crescenti, preoccupanti e probabilmente vere, sostengono che il processo di privatizzazione, che sarebbe possibile nel territorio romano e nella città di Roma, porterebbe il controllo dell'ACEA nelle mani del più grande costruttore edile dell'area. L'azienda di Caltagirone, già arbitra del piano regolatore, degli equilibri territoriali, della massa infinita di costruzioni edilizie che verranno riversate e continueranno ad essere riversate sul territorio romano, di tutti quegli equilibri che stanno tra la politica e gli affari, potrebbe entrare in possesso anche del soggetto che controlla l'acqua.

Così come vi è il monopolista dei mezzi di comunicazione, che può comandare il vertice del potere politico, cosa che nessun altro Paese democratico avrebbe mai accettato - solo a noi è capitata questa disgrazia

provvedimento in esame presenta un duplice ambito di rilevanza sia sul piano istituzionale, in rapporto all'adozione di un nuovo approccio di adeguamento del diritto interno a quello comunitario, sia per gli interventi settoriali disciplinati dall'articolato. Il nostro Paese si è da sempre distinto per l'alto numero delle infrazioni comunitarie, per motivi legati anche alla complessità del procedimento legislativo italiano, incentrato - com'è noto - sul bicameralismo perfetto. Questa lentezza del nostro Paese nell'adeguamento alla normativa comunitaria ha prodotto negli ultimi anni rilevanti conseguenze di tipo economico, essendo stata riconosciuta alla Corte di giustizia europea la facoltà di applicare sanzioni finanziarie al momento della constatazione dell'infrazione. Tale evoluzione nel rapporto tra il diritto comunitario e quello interno impone una più netta assunzione di responsabilità, finalizzata ad adottare - anche in chiave preventiva - tempestivi correttivi. È forse superfluo ricordare al riguardo che attualmente risultano aperte 16 procedure d'infrazione ex articolo 228 del Trattato CE, alcune delle quali sono oggetto di specifiche disposizioni negli articoli del presente decreto. Appare chiaro che si è presa coscienza del fatto che la massa delle norme del diritto comunitario che necessitano di essere trasposte nella nostra legislazione è tale che anche lo strumento della decretazione d'urgenza, previsto dall'articolo 10 della legge Buttiglione,

Accanto a queste considerazioni generali di rilievo istituzionale, è innegabile come il provvedimento presenti specifici profili d'interesse in rapporto alle tematiche affrontate nelle discipline di settore. Si tratta di interventi trasversali ai diversi settori delle politiche pubbliche, dai trasporti al trattamento dei rifiuti, dai regimi fiscali ai servizi pubblici locali.

Con riferimento all'articolo 15, è noto - perché è già stato detto - che secondo il parere della 14ª Commissione sarebbe stato preferibile trattare questa materia in un provvedimento a parte. Bisogna però riconoscere che il dibattito su questo tema è stato abbastanza ampio e che anche durante la discussione in Aula sono state apportate alcune opportune modifiche. È noto che negli ultimi otto anni sono state approvate ben quattro riforme dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Il contesto di riferimento, tuttavia, è stato modificato di poco, se si escludono alcuni importanti processi di aggregazione aziendale del Nord. Rispetto a quest'articolato percorso di riforme, l'articolo 15 del provvedimento in votazione prosegue la privatizzazione iniziata al principio degli anni '90. In realtà, la privatizzazione e la liberalizzazione dei servizi pubblici locali non sempre sono state accompagnate da una discesa dei costi per l'utenza e dall'effettivo soddisfacimento dei cittadini. Le tanto discusse municipalizzate, ora trasformate in gestioni *in* *house*, spesso hanno dimostrato il raggiungimento di livelli di servizio, di efficienza e di economicità difficilmente raggiungibili con una gestione esternalizzata a privati. Inoltre, tali società *in* *house* hanno spesso raggiunto esperienze operative e modelli d'impresa che occorre sostenere, fortificare e far crescere, perché sono quelli che potranno rappresentare il nostro Paese all'estero, all'apertura del mercato europeo; altrimenti, rischiamo di consegnare i nostri servizi alle imprese straniere, vista la necessità di applicare le norme comunitarie sugli appalti e sulla libera concorrenza nel contesto europeo. Sulla base di queste premesse, la Lega Nord ha da sempre sostenuto la possibilità per i Comuni di scegliere liberamente la forma più appropriata di gestione dei propri servizi pubblici locali, di evitare le gare per le realtà territoriali minori e i piccoli Comuni, di promuovere la crescita delle nostre imprese ex municipalizzate, assegnando loro congrui periodi transitori che permettano loro di diventare competitive sul mercato europeo. La riforma dei servizi pubblici locali, introdotta con l'articolo 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, ha cercato di mettere d'accordo le svariate posizioni delle componenti politiche. Non si può tuttavia mancare di evidenziare come l'applicazione marginale degli affidamenti *in* prevista da tale riforma rischi di diventare isolata nell'ambito comunitario, che invece consente un ampio accesso a questa formula gestionale, se correttamente applicata.

Il nucleo centrale della riforma coincide, in particolare, con la disciplina del partenariato pubblico privato, alla pari della procedura competitiva per l'affidamento del servizio, a condizione che con la stessa gara si scelga il socio e si attribuiscano i compiti operativi connessi alla gestione del servizio; come previsto dall'ultimo orientamento della Comunità europea, del resto. La novità, solo italiana, è l'inserimento di un limite alla partecipazione privata nella società, non inferiore al 40 per cento. Tale limite da una parte renderebbe appetibile la partecipazione privata nella società, ritagliando un mercato utile per le imprese locali e minori. La gestione *in* *house* è rimasta per particolari situazioni territoriali, molto estese ed indefinite; si ricorda che anche questa restrizione è una scelta tutta italiana, perché l'Unione europea riconosce a tutti la possibilità della gestione *in* Al riguardo, tutti convergono nell'opinione che fino ad oggi l'Antitrust abbia adottato criteri estremamente rigidi per vagliare l'esistenza delle condizioni per la costituzione delle strutture *in* *house*, con la conseguenza di "bocciare" letteralmente, sempre, la costituzione di nuove società. Per questo motivo, uno degli emendamenti della Lega Nord approvati in Commissione, in coerenza con tutto il percorso compiuto dalla Lega nel lungo dibattito parlamentare su servizi pubblici locali, affida al regolamento, invece che all'Antitrust, l'individuazione delle soglie minime al di sotto delle quali non diventa necessario l'intervento della stessa Antitrust. Grazie a questa e alle altre modifiche apportate in Commissione all'originaria formulazione dell'articolo 15, ci auguriamo che la nuova disciplina possa effettivamente contribuire a salvaguardare sia le istanze di concorrenzialità del mercato, sia le esigenze - che in questo settore appaiono prioritarie - di tutela degli interessi pubblici nella regolazione dei servizi. Con riferimento all'articolo 16, voglio evidenziare come tale disposizione sia finalizzata a delineare un quadro normativo certo ed univoco attraverso cui viene disciplinato, e quindi tutelato, il *made in Italy*. L'obiettivo è quello di evitare che le attuali incertezze del nostro ordinamento in materia possano favorire l'ingresso nel Paese di prodotti contraffatti, spesso provenienti dai Paesi del Sud Est asiatico, a danno delle imprese nazionali. Di primario interesse, in particolare, la disposizione che consente di classificare come *made* *in* *Italy* solo i prodotti o le merci il cui disegno, progettazione, lavorazione e confezionamento siano compiuti interamente sul territorio italiano. Chiunque fa uso di un'indicazione di vendita fallace, allo scopo di ingannare il consumatore sull'acquisto di prodotti che, pur essendo etichettati *made* *in* *Italy*, non sono stati interamente realizzati sul territorio italiano, sarà punito con la reclusione fino a due anni e la multa fino a 20.000 euro. Questa previsione accoglie istanze da tempo avvertite dalla Lega Nord e tradotte anche in apposite iniziative legislative, particolarmente urgenti in un periodo di crisi economica come quello attuale. La concorrenza proveniente dai Paesi terzi, con particolare riguardo all'Est asiatico, impone infatti l'azione di misure correttive, che, senza infrangere il principio della libera circolazione delle merci, sappiano promuovere una nuova immagine della produzione nazionale, conforme a standard di qualità garantiti anche attraverso la tracciatura dell'intero percorso produttivo. È opportuno evidenziare come questo intervento sia destinato a favorire non solo le grandi imprese, che rendono famoso il nome dell'Italia all'estero, ma anche l'importante e spesso sottovalutato comparto delle piccole e medie imprese che, specialmente in alcuni settori (come il tessile, la concia, il mobile), rappresentano l'autentica speranza per il rilancio dell'economia nazionale. Inoltre, la misura in esame è destinata ad offrire risposte all'esigenza di un'effettiva trasparenza in merito al luogo di origine delle materie e della produzione. l'articolo 16 predispone strumenti fondamentali per combattere il fenomeno della contraffazione attraverso l'adozione di un sistema di etichettatura di origine dei prodotti che tuteli imprese e consumatori. Nel complesso, anche a considerare l'atipicità dell'*iter* legislativo seguito dal provvedimento in esame e l'esigenza di ricondurne le sorti alla competenza della 14ª Commissione

già approvata alla Camera ed assegnata al Senato), intendo riconoscere il lavoro svolto dalla 1ª Commissione e dal relatore sul decreto-legge

Signor Presidente, onorevoli colleghi, alcune settimane fa la presidente del nostro Gruppo, Anna Finocchiaro, insieme ai vice capigruppo Zanda e Latorre e a molti senatori del Partito Democratico, ha presentato una mozione che spero possa essere discussa prima possibile. Essa si occupa di un delicato aspetto della vita democratica del nostro Paese. Si esprime infatti la preoccupazione che siamo di fronte a una modifica della Costituzione materiale così profonda da farci ritenere, con assoluta serenità,

e in primo luogo tra il potere legislativo, che spetta al Parlamento, il potere esecutivo, attribuito al Governo, e la funzione giurisdizionale, affidata alla magistratura. Colleghi, la vicenda parlamentare che si conclude questa sera in questo ramo

la Costituzione materiale e di come il potere legislativo sia soltanto formalmente ascritto alla responsabilità del Parlamento. Innanzitutto, si tratta di un decreto‑legge che reca nel titolo una denominazione estremamente circoscritta: si parla delle violazioni delle direttive comunitarie e delle possibilità di adeguare la legislazione italiana ad obblighi comunitari. In realtà, si tratta di una materia che, di fatto, già nel decreto-legge si presenta Si parla ormai chiaramente, spesso anche per riferirsi a tale provvedimento, di un vero e proprio decreto *omnibus*, in cui ci sono le più varie e disparate

Ora, il fatto che una riforma di questa ampiezza e di questa profondità venga attuata senza avere la possibilità di svolgere, per esempio, un'approfondita discussione con il mondo degli enti locali, con le Regioni, con le Province, se non in una fugacissima e molto compressa audizione,

che, in materia di servizi pubblici locali, erano già stati presentati in Parlamento alcuni disegni di legge e che l'esame parlamentare nella Commissione affari costituzionali era già iniziato. Per un dovere di cortesia istituzionale noi abbiamo fermato l'esame in attesa che il Governo, che aveva preannunciato un disegno di legge, lo presentasse.

con il solo obiettivo di ottenere l'effetto annuncio di dire che il Governo, finalmente, dopo tanti anni ha fatto la riforma dei servizi pubblici locali. Si realizza una presunta privatizzazione assai poco coraggiosa.

con il quale si passa dall'*opt-out* all'*opt-in.* Come ho già detto poco fa, nel corso dell'intervento con cui abbiamo motivato il nostro voto contrario: è inutile che il relatore

Questa vicenda parlamentare che oggi si conclude è una brutta pagina del lavoro parlamentare di questa legislatura. E' un ulteriore gradino che scendiamo nella trasformazione del nostro sistema parlamentare, in cui al Parlamento viene sottratta nella sostanza e non nella forma la funzione legislativa. Si tratta di un decreto diventato un'arlecchinata, con pezze di tutti i colori; è una brutta pagina, perché una riforma che avremmo potuto fare con ben altro coraggio, invece, ha sostanzialmente partorito un topolino! Nessun serio intervento riformatore. Si tratta di una brutta pagina perché queste riforme nella prassi parlamentare -basta andare a vedere come avviene - non sono più scritte dal Parlamento o dalle Commissioni, ma dagli uffici legislativi dei Ministeri, che sono coloro i quali non solo presentano le norme del decreto-legge, ma poi presentano anche gli emendamenti a firma del relatore e di altri.

il nostro Paese si trasforma sempre di più in una giungla in cui più forte, il più furbo, il più spericolato riesce ad avere una condizione di vantaggio. Presidente, per queste ragioni, i senatori del Partito Democratico con profonda convinzione voteranno no al disegno di legge di conversione del decreto-legge che oggi abbiamo esaminato.

Presidente, colleghi, non è facile prendere la parola in conclusione di un dibattito così ampio. Sono state ore e ore di interessante discussione, nell'ambito della quale ciascuno ha evidenziato le proprie posizioni, sia politiche sia giuridiche. servirebbe a ribadire come non ci sia espropriazione del Parlamento nell'attività legislativa; è un concetto che ho già espresso quando ho illustrato il mio contrasto alla questione pregiudiziale Bisogna dire che il nostro Parlamento, ed il Senato *in primis*, lavora intensamente, e bene. In Commissione questo provvedimento è stato discusso a lungo. Ci sono stati apporti, anche dell'opposizione, estremamente interessanti, e si è arrivati in Aula per mettere in essere questa ampia discussione sul testo e sugli emendamenti. Cosa si vuol dire? Si vuol dire che non possiamo usare concetti pesanti come quelli espressi in questi ultimi interventi. Quando diciamo che la Costituzione materiale ha superato la Costituzione scritta, diciamo delle cose che in parte appartengono alla propaganda ed in parte non tengono conto della evoluzione legislativa quotidiana, sia a livello di produzione governativa sia soprattutto a livello di convalida parlamentare. Noi sappiamo quali e quante siano le esigenze di immediatezza negli interventi ed allora comprendiamo come il ricorso ai decreti-legge sia necessario. D'altro canto, non voglio sottolineare l'argomento, ma le vostre critiche sono quelle che noi facevamo nei due anni passati di opposizione, nella XV legislatura, direi quasi in termini precisi, di comparazione esatta. Anche noi ci lamentavamo del troppo frequente ricorso ai decreti-legge; anche noi criticavamo un determinato modo di affrontare gli emendamenti nei decreti-legge, di inserire emendamenti in parte poco pertinenti, in parte talmente importanti che avrebbero richiesto una discussione in separati provvedimenti legislativi.

Non a caso nei progetti di riforma costituzionale è prevista anche la riforma dell'articolo 77 della Costituzione nei termini che ciascuno potrà vedere andando a leggere quei testi. Perché? Perché in tempi di globalizzazione il procedimento legislativo deve essere forzatamente reso celere. celere. È facile dire che abbiamo già approvato quattro riforme dei servizi pubblici essenziali e che adesso ne abbiamo approvata un'altra; dovevamo però approvarla con la legge che si stava cominciando a discutere in Parlamento: invece si è intervenuti con un emendamento ad un decreto‑legge.

la riforma attuale in tempi brevi, pur nell'ampiezza della discussione. Ma perché? Lo ha spiegato così bene la presidente Boldi: siamo in un momento nel quale con il Trattato di Lisbona cambierà completamente il nostro modo di legiferare. Già oggi gli interventi europei sono talmente pregnanti ci costringono a prendere atto di una situazione nuova che importa velocizzazione del procedimento legislativo. Probabilmente la legge sui servizi pubblici essenziali, se discussa con calma in Commissione, avrebbe necessitato di mesi, e non c'era la possibilità di aspettare tanto. Questo è il punto. Quindi, attenzione con le critiche, perché, ripeto, sono le stesse critiche che abbiamo sviluppato nella XV legislatura nei vostri confronti, e anche le altre volte quando siamo stati all'opposizione. Oggi come oggi bisogna dire che si è risolto questo problema dei servizi pubblici essenziali in termini ampiamente accettabili, e di questo siamo soddisfatti, in una linea europea, (come ancora ricordava la presidente Boldi) di cambiamento della situazione rispetto, per esempio, alle gestioni delle municipalizzate e più ampiamente delle gestioni *in house*, perché si torna ad una liberalizzazione che è quella che oggi vuole l'Europa. Non è che potremmo chiuderci dicendo che le nostre ottime - che poi non lo sono, o perlomeno ce ne sono pochissime - municipalizzate fanno parte del nostro patrimonio storico e ci teniamo quelle,

fra l'Europa e l'Italia; in parte, in un'ottica di obblighi comunitari percepiti e comunque reali, tipo il discorso dei servizi pubblici essenziali nei suoi sviluppi immediatamente futuri, che ci hanno portato a provvedere.

bravo umorista che descrive la guerra dell'acqua come la sconfitta del pubblico; ma è soltanto un bel libro umoristico, che in alcun modo può dipingere una realtà, perché questa realtà non esiste. L'acqua in Italia è

Quindi l'intervento del collega Pardi è stato catastrofista, e non possiamo in alcun modo accettarlo; accettare le critiche al modo di legiferare, quando non hanno un vero valore se non polemico. Il senatore Bianco, al quale va tutto il mio rispetto e, se lui mi permette, anche la mia amicizia, dice che le leggi le scrivono nei Ministeri, le passano ai Ministri e le fanno firmare ai parlamentari. Non è così!

di ordine pubblico, sicurezza, riforme costituzionali e quant'altro, e quando affrontiamo provvedimenti relativi a materie tecniche, diverse dalle nostre, ci vediamo costretti ad uno sforzo ulteriore che comunque facciamo volentieri,

solo pochi attimi per richiamare l'attenzione sul voto che stiamo per esprimere. Il senatore Di Girolamo, essendo stato eletto sindaco della sua città, si dimette da senatore: è un gesto di sensibilità e di responsabilità. Vorrei richiamare però l'attenzione sul fatto che il senatore Di Girolamo avrebbe potuto tranquillamente non dimettersi, come in altri casi è successo: a partire dall'elezione dell'onorevole Cammarata a sindaco di Palermo, si è instaurata una giurisprudenza ovviamente perfettamente legittima dal punto di vista della legge, ma credo più discutibile dal punto di vista del costume politico - che induce sindaci e presidenti di Provincia a cumulare la loro responsabilità amministrativa con il mandato parlamentare. Vorrei ricordare che, nella cosiddetta prima Repubblica, in 47 casi si ritenne sufficiente una prassi per imporre le dimissioni di sindaci e presidenti di Provincia: lo dico non per intonare lo stucchevole ritornello sul «si stava meglio meglio quando si stava peggio», ma per mettere noi stessi sull'avviso di una deriva che abbiamo preso, che comporta oggi qualche piccolo vantaggio per le persone, ma comporterà sicuramente domani un grande danno per le istituzioni e per la credibilità di tutti noi. Con i senatori Augello, D'Alia e Sanna, abbiamo presentato una proposta *multipartisan* che stabilisce un regime di incompatibilità più rigoroso e che dovrebbe metterci al riparo da questa situazione di doppio incarico, per così dire. Richiamo l'attenzione della Presidenza del Senato e della Conferenza dei Capigruppo sull'urgenza di calendarizzare questa proposta, poiché essa non contiene nessuna guerra alla «casta», ma credo che comporti la pace con il buonsenso, e mi auguro che quella pace la faremo presto.

i senatori che intendono astenersi premeranno il tasto bianco a sinistra. Poiché si tratta di una votazione a scrutinio segreto, qualunque sia la scelta di voto effettuata, la luce che si accenderà sarà ovviamente di colore neutro. Dichiaro aperta la votazione. *(Segue

Per consentire alla Giunta delle elezioni di procedere all'accertamento del candidato subentrante al senatore dimissionario, autorizzo la Giunta delle elezioni a convocarsi sin d'ora nell'adiacente Sala Pannini.

Signor Presidente, colleghi, la prospettiva di finanza pubblica delineata nei documenti di bilancio per il prossimo triennio registra il superamento del punto di minimo di una crisi economica e finanziaria molto forte, e i primi sintomi di una ripresa segnalata anche da autorevoli istituzioni internazionali. In un contesto generale caratterizzato da elevata incertezza sulle prospettive economiche, il Governo in questi mesi ha scelto una forte prudenza per evitare effetti indesiderati di retroazione di manovre espansive sulle variabili macroeconomiche. Chiuso l'esercizio 2009, non è stato ritenuto opportuno operare una correzione sui conti pubblici del 2010. Il percorso di risanamento delle finanze pubbliche riprenderà nel 2011, quando la fase ciclica sarà più favorevole, e proseguirà nel 2012 e nel 2013. L'opposizione, anche nel confronto in Commissione, confuta tale impostazione, proponendo politiche espansive per uscire prima dalla crisi. Ma tale opzione non considera, a nostro modo di vedere, compiutamente i rischi di peggiorare in modo significativo il *deficit* per un Paese come l'Italia che ha uno dei debiti pubblici più elevati in rapporto al PIL. D'altro canto, perché non sfruttare questo periodo per analizzare e individuare soluzioni efficaci per ridurre la spesa a partire dal 2011 e per il triennio successivo? I quadri riassuntivi del bilancio e gli allegati al disegno di legge finanziaria forniscono il quadro di quanto detto. Sul conto consolidato della pubblica amministrazione, la manovra in esame non produce effetti per il triennio. In termini di amministrazioni centrali (ossia il bilancio dello Stato) il quadro riepilogativo del bilancio 2010, posto a confronto con il bilancio assestato del 2009, mostra un miglioramento del*deficit* (saldo netto da finanziare) di circa 8,5 miliardi. Tale miglioramento è il risultato di una riduzione delle spese correnti di 2 miliardi e delle spese in conto capitale di oltre 8 miliardi, da un lato, e, dall'altro, della riduzione delle entrate per circa 0,7 miliardi e di un aumento della spesa per interessi di oltre un miliardo. Sul 2010, poi, l'effetto delle tabelle della legge finanziaria determina un peggioramento del saldo di circa 1,3 miliardi. In altre parole, le tabelle alla legge finanziaria producono effetti espansivi rispetto al saldo di bilancio a legislazione vigente, ma il saldo finale per il 2010 è migliore rispetto a quello risultante dall'assestamento 2009: rispetto ai 69,7 miliardi del 2009, le previsioni per il bilancio dello Stato, integrato con il disegno di legge finanziaria, portano a un saldo netto da finanziare per circa 62,4 miliardi. La sfida, colleghi, per i prossimi anni, una volta che l'economia sarà tornata al livello di stabilità, è riprendere con maggior vigore il cammino di risanamento dei conti pubblici, tenuto conto del deterioramento conseguente alla crisi economica e finanziaria. Se l'obiettivo è quello di ridurre, a partire dal 2011, le spese per migliorare i conti pubblici, ci chiediamo quali strumenti si possono mettere in campo, quali informazioni possiamo desumere già dal bilancio per individuare spazi idonei a ridurre le spese per il futuro. Come è noto, il tema è particolarmente rilevante, tenuto tenuto conto che, come segnalato dalla Banca d'Italia durante le audizioni, il raggiungimento dell'obiettivo indicato per il disavanzo del 2013, vale a dire il 2,2 per cento richiede che le spese correnti primarie si riducano in termini reali in media di quasi l'1 per cento all'anno nel periodo 2010‑2013, assumendo ovviamente che il prodotto cresca del 2 per cento triennio, che siano confermati i livelli tendenziali delle entrate e degli interessi e che le spese in conto capitale restino stabili in rapporto al PIL sul valore del 2010. Si tenga poi conto che nell'ultimo decennio 1998-2008 le spese correnti primarie in termini reali sono aumentate in media del 2,1 per cento spiega quanto sia importante e delicata la sfida di cui abbiamo parlato. Strumenti per verificare quanto sia rigida la spesa e quali spazi vi siano effettivamente per ridurla, in parte sono contenuti anche nel disegno di legge di bilancio stesso. La riclassificazione per missioni e programmi è un primo aspetto che descrive la capacità redistributiva del bilancio. Infatti la ripartizione per missioni della spesa del bilancio per l'anno 2010 evidenzia come le voci di spesa con una rilevanza superiore al 5 per cento del siano le seguenti missioni: il debito pubblico (si tratta degli interessi, ossia dell'onere e dei rimborsi del debito), che è pari al 42,7 del totale della spesa; relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, pari al 14,5 per cento; politiche previdenziali, pari al 9,7 per cento; politiche economiche e finanziarie, pari all'8 per cento; istruzione scolastica, per cento. Queste indicazioni danno un quadro sommario della decisione di spesa del Parlamento, nella misura in cui gli interessi e i rimborsi sul debito rappresentano un elemento estraneo alle scelte del Parlamento, e come tale deve essere considerato come un dato del problema. Al pari, i trasferimenti alle altre amministrazioni pubbliche sono elementi di rigidità, derivanti dal fatto che in un sistema di governo multilivello sussiste ancora una rilevante quota di trasferimenti dal governo centrale ai livelli decentrati; eliminando eliminando infatti la missione del debito, i trasferimenti alle amministrazioni e il programma delle regolazioni debitorie, le missioni che hanno una consistenza percentuale superiore al 5 per cento del totale della spesa sono l'istruzione scolastica, l'Italia in Europa e nel mondo, la difesa e la sicurezza del territorio, i fondi da ripartire, le politiche previdenziali, l'ordine pubblico e la giustizia. Si può far riferimento alle tabelle che abbiamo messo in distribuzione a corredo della possibile verificare se e in che misura il bilancio dello Stato ha natura di trasferimento e quante risorse invece rimangono, signor Presidente, nella competenza dei Ministeri per le politiche pubbliche dello Stato centrale. A tal riguardo, la spesa complessiva delle missioni per l'anno 2010 è pari a 792,7 miliardi di euro, mentre la spesa complessiva al netto della missione del debito pubblico, dei trasferimenti e delle regolazioni debitorie, scende a 180,6 miliardi, pari cioè al 23 per cento. Da ciò si desume che il 77 per cento circa delle spese del bilancio dello Stato è composto da spese esogene (gli interessi e il rimborso del debito) o da trasferimenti ad altre amministrazioni pubbliche e dunque che il bilancio dello Stato per oltre i tre quarti è fatto di trasferimenti. La classificazione economica del bilancio ci fornisce indicazioni ulteriori sui margini di flessibilità dello stesso; infatti dai dati indicati si rileva che 91,6 miliardi dei 180 sono spese il personale, difficilmente rimodulabili nel medio termine. L'analisi dei redditi da lavoro dipendente classificati per missione evidenza che il 44 per cento dei 91 milioni è destinato all'istruzione scolastica. L'ammontare dei consumi intermedi, voce sulla quale si è intervenuti in passato per migliorare i conti pubblici, è pari nel 2010 a circa 8 miliardi di euro. Le risorse proprie dell'Unione europea a carico del bilancio dello Stato sono pari a 17 miliardi Le risorse correnti destinate ad attuare le politiche pubbliche attraverso il bilancio per trasferimenti alle famiglie sono pari soltanto a 3,8 miliardi per il 2010, mentre quelli per trasferimenti alle imprese sono pari a 4,2 miliardi. Se si tiene conto anche delle agevolazioni fiscali riconosciute come minori entrate per le famiglie e le imprese, agli importi precedenti si aggiungono circa 6 miliardi. Da quanto detto sembrerebbe emergere, con tutte le cautele derivanti da un'analisi limitata al bilancio dello Stato, che gli spazi per politiche redistributive operate mediante il bilancio dello Stato non siano molto ampi nel breve periodo. Non è quindi un caso che il confronto sulle opzioni di politica economica da adottare durante la sessione di bilancio svolto tra la maggioranza, il Governo e l'opposizione, abbia riguardato lo sgravio IRAP sul monte salari per le piccole e medie imprese, coperto attraverso la soppressione dei trasferimenti in conto corrente ed in conto capitale a fondo perduto alle imprese, per un importo di circa 6 miliardi. Con ciò confermando l'analisi sopra svolta che le scelte redistributive operate nel breve termine possono interessare soltanto le voci dei trasferimenti alle imprese ed alle famiglie per importi inferiori ai 10 miliardi rispetto ad un volume di spese molto più elevato ma anche poco modulabile nell'arco di un anno. A mio avviso, è da considerare con interesse il dibattito aperto sull'opportunità di ridurre le imposte a beneficio di tutti piuttosto che mantenere contributi a singole imprese. Nel medio e lungo termine, a livello di pubbliche amministrazioni, invece, molto si può attendere anche dal federalismo fiscale, in quanto può determinare un incentivo a spendere meglio per aumentare i margini di intervento della politica. Per quanto riguarda il bilancio dello Stato, nonostante il quadro delineato, ulteriori margini di intervento possono derivare dalla revisione della spesa. A tal riguardo, occorre segnalare una novità recente di grande ausilio per il Parlamento. Mi riferisco al Rapporto sulla spesa delle amministrazioni centrali dello Stato per l'anno 2009 elaborato dalla Ragioneria generale dello Stato e non ancora trasmesso al Parlamento. Si tratta di un copioso lavoro di analisi per comprendere meglio i meccanismi di formazione della spesa. Soltanto conoscendo tali meccanismi è possibile capire come ridurre la spesa, inclusa quella di personale che abbiamo visto quanto pesi, aumentando la produttività e senza necessariamente ridurre la qualità dei servizi pubblici. Occorre segnalare che nel dibattito svolto nelle Commissioni di merito, ad eccezione della Commissione istruzione, gli elementi contenuti nel Rapporto non sono stati richiamati. Non si è ancora instaurato un circolo virtuoso che vede da un lato il ruolo della Ragioneria di supporto ai Ministeri per conoscere meglio la spesa e, dall'altro, il ruolo di controllo del Parlamento che, utilizzando le stesse analisi, chiama i dirigenti generali a spiegare le ragioni di eventuali spese che non appaiono efficienti. Si tratta ovviamente di un processo graduale. L'auspicio è che tali strumenti conoscitivi vengano affinati e impiegati nei prossimi esercizi. alcune questioni metodologiche. Vi sono alcuni aspetti da segnalare dell'attuazione della riclassificazione del bilancio per missioni e programmi rispetto al precedente bilancio amministrativo, che trovano immediato riscontro nel dibattito sulla riforma dei documenti di bilancio in esame presso l'altro ramo del Parlamento. Il nuovo bilancio rappresenta indubbiamente un miglioramento del precedente. Consente di capire meglio come vengono destinate le risorse; sono stati elaborati per ogni programma alcuni indicatori di *performance*, al fine di spiegare in modo molto dettagliato l'articolazione e gli effetti delle politiche pubbliche operate con il bilancio. è una valutazione preliminare di questa esperienza. Cosa misurano gli indicatori scelti dalle amministrazioni? Secondo quanto indicato dal lavoro «Una analisi degli indicatori di di *performance* nelle note preliminari 2008-2009» elaborato dalla Ragioneria generale dello Stato, emerge che «una quota piuttosto elevata di indicatori individuati dalle amministrazioni sono poco chiari», oppure che «il valore-obiettivo non è coerente con l'indicatore utilizzato per misurarlo». Ovviamente tra il 2008 ed il 2009 vi sono stati progressi nelle schede a corredo del bilancio, in termini di completezza dell'informazione fornita, ma il processo è in corso e sussistono ampi margini di miglioramento. È auspicabile che le Commissioni di merito «si approprino» in futuro delle proprie missioni e si impegnino a verificare l'adeguatezza degli indicatori di *performance* - a memoria, senatore Morando - a descrivere l'effetto delle politiche pubbliche al fine di svolgere il controllo sull'efficacia dei programmi.

durante l'esame in Commissione del disegno di legge di bilancio, sono stati approvati emendamenti di importi poco significativi, che non alterano nella sostanza l'originaria distribuzione delle risorse tra le varie voci. La Commissione ed il Governo hanno ritenuto inopportuno in questa fase approvare un emendamento già approvato durante l'esame del bilancio in sede consultiva dalla Commissione giustizia. L'opposizione ha lamentato che nel bilancio in esame vi sono, tra l'altro, tagli al Fondo per l'occupazione, ai fondi per la costruzione di nuovi istituti penitenziari, al funzionamento della giustizia, per citarne alcuni. Alcuni rilievi sul settore dell'istruzione sono stati parzialmente accolti approvando emendamenti in Commissione. l'ottica corretta è a nostro avviso quella di concentrare l'attenzione del dibattito sull'impostazione generale del bilancio, anziché su singoli aspetti. La decisione di spesa assunta con il bilancio presuppone nel complesso un miglioramento dei saldi, lo si è già detto. A ciò si aggiunga che alcune missioni hanno determinato un aumento di spesa: la missione debito pubblico ha subito un incremento di 45 miliardi di euro, quella per i trasferimenti alle autonomie territoriali di 1,7 miliardi. In questo quadro generale, di una scelta complessiva di miglioramento dei saldi, e di alcune spese che inevitabilmente hanno richiesto maggiori risorse, è evidente che alcune missioni hanno dovuto subire dei tagli. A fronte di ciò, sono state incrementate le risorse per lo sviluppo ed il riequilibrio territoriale e per le infrastrutture. In altri termini, la visione micro-analitica focalizzata sul singolo taglio ad un settore specifico o ad un ad un fondo particolare, non appare il tema proprio del dibattito sulla decisione di bilancio. Sarebbe preferibile che tali dettagli venissero discussi nelle Commissioni di merito. A tal riguardo, sarebbe utile una riflessione comune sulle procedure di analisi del bilancio conseguenti alla riclassificazione dello stesso per missioni e programmi, chiedendosi se ha senso ancora mantenere l'attuale procedura di discussione del bilancio che pospone l'esame della Commissione bilancio dopo quello delle Commissioni di merito. Per concludere, nel breve periodo gli ambiti di manovra per svolgere politiche redistributive non sono molto ampi, e questo è un dato che prescinde da qualsiasi valutazione politica, di parte o di schieramento. Per questo siamo tutti chiamati ad accogliere la sfida di lavorare insieme nelle Commissioni di merito per capire i meccanismi di formazione della spesa e per tagliare gli interventi privi di ogni effetto sulle politiche pubbliche. Ciò consentirà, *in primis*, di risanare i conti pubblici tagliando la spesa inefficiente e, successivamente, di avere spazi più ampi per fare le politiche richieste dai cittadini e dalle imprese. Soltanto attraverso questo lavoro puntuale e metodico possiamo riappropriarci di margini più ampi di manovra per «fare le politiche pubbliche»; altrimenti siamo condannati a relegare le grandi scelte di politica economica a spazi limitati per aiutare le imprese a diventare più competitive le famiglie a creare più ricchezza. Se non si realizza tale obiettivo sarà difficile immaginare di aumentare il benessere del Paese. Si impone dunque che le Commissioni di merito esaminino sistematicamente, durante l'anno, l'efficacia della spesa nei settori di competenza in un confronto virtuoso con i dirigenti responsabili della spesa medesima. Il bilancio ora ci consente di analizzare tutti i microinterventi sottostanti ai programmi e alle missioni. Questo lavoro non può essere limitato alle due sedute dedicate all'esame del bilancio nelle Commissioni di merito una volta l'anno. Questo è un lavoro che richiede una costanza durante tutto l'anno e che nell'esame del rendiconto trova poi la sede idonea per misurare i risultati ottenuti o eventuali scostamenti. il contesto politico attuale ed i vincoli economico-finanziari, senza dividerci tra i rigoristi e quelli del partito della spesa, impongono al Parlamento di concentrare le proprie funzioni e attività sul tema del controllo della spesa e della sua qualificazione.

Luigi Sturzo nel 1958 sosteneva che l'immoralità si corregge non con le prediche, ma con un'amministrazione capace di premiare il merito.

il disegno di legge finanziaria per il 2010 vede confermata l'impostazione semplificata già presentata nella manovra dello scorso anno, sia in quanto a contenuto normativo, sia in termini di effetti sui saldi di finanza pubblica. Anche per il 2010 viene infatti proposta una finanziaria snella, che si articola in soli tre articoli, il cui contenuto è essenzialmente riconducibile a quello considerato più tipico della legge. Le norme contenute nel provvedimento in esame si limitano infatti, come di consueto, a fissare gli obiettivi dei saldi di bilancio, a disporre la proroga di norme di carattere tributario recanti regimi agevolati, a definire l'importo delle risorse destinate ai rinnovi contrattuali nonché l'importo dei trasferimenti destinati agli enti previdenziali e, infine, a stabilire l'importo da iscrivere nelle tabelle allegate. altresì che anche la manovra finanziaria per il triennio 2010-2012, pur essendo incentrata sui due tradizionali strumenti legislativi, il disegno di bilancio a legislazione vigente e il disegno di legge finanziaria, ha visto anticipati buona parte dei suoi effetti dalle disposizioni previste dal decreto-legge n. 112 del 2008, con cui si è provveduto alla definizione dello scenario finanziario per il triennio 2009-2011.

strettamente attinenti al suo contenuto tipico, con l'esclusione di disposizioni finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, nonché di carattere ordinamentale, microsettoriale e localistico. A ben vedere, le disposizioni contenute nel provvedimento confermano pertanto, nel complesso, come già segnalato lo scorso anno, un assetto della decisione di bilancio più simile a quello vigente prima della legge di riforma del 1999, la quale, raggiunto il traguardo dell'ingresso nell'euro, dispose, tra le altre cose, un ampliamento del contenuto cosiddetto proprio e sino ad allora maggiormente tipizzato della legge finanziaria. La conferma del ridimensionamento del contenuto della legge finanziaria rispetto alla prassi seguita negli anni più recenti è accompagnata da una valorizzazione del contenuto decisionale del bilancio dello Stato, stante la possibilità nella legge di bilancio - anche per il 2010, dopo l'avvio di una fase sperimentale già attivata per il 2009 di rimodulare, tra i programmi, le dotazioni finanziarie di ciascuna missione, ivi incluse le risorse derivanti da autorizzazioni legislative di spesa. Nel dettaglio, per quanto concerne gli effetti sui saldi di finanza pubblica, il disegno di legge finanziaria per il 2010 non comporta effetti correttivi in termini di indebitamento netto del conto economico delle amministrazioni pubbliche, la cui incidenza sul PIL rimane pertanto fissata per il triennio 2010-2012 nei valori indicati dalla Nota di aggiornamento al DPEF. Venendo al contenuto, l'articolo 1 reca la consueta fissazione del livello massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 2010, al netto delle regolazioni debitorie, in 63.000 milioni di euro e il livello massimo del ricorso al mercato per lo stesso periodo in 286.000 milioni di euro. L'articolo 2, dal comma 1 al comma 4, reca invece disposizioni in materia di regolazione di trasferimenti a carico del bilancio dello Stato per il riequilibrio delle gestioni previdenziali, mentre al comma 5 si stabilisce che il termine per la rilevazione della media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro ai fini della determinazione della retribuzione media convenzionale da porre a base per i trattamenti pensionistici e per il calcolo dei contributi degli operai agricoli a tempo determinato sia lo stesso di quello previsto per gli operai a tempo indeterminato. Inoltre, l'articolo 2, comma 7, dispone la modifica del comma 17 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2008, prorogando per l'anno 2012 le agevolazioni contenute nel medesimo comma in materia di imposte dirette in tema di spese sostenute per ristrutturazioni immobiliari, mentre il comma 8 modifica il comma 18 della legge finanziaria per il 2008, prorogando agli anni 2012 e successivi l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata al 10 per cento nel medesimo settore. Ai commi da 9 a 11 del medesimo articolo, nelle more della definizione degli stanziamenti destinati ai rinnovi contrattuali, sono invece indicate le autorizzazioni di spesa connesse al riconoscimento della prevista indennità di vacanza contrattuale per i dipendenti pubblici, mentre ai successivi commi 12-16 si prevedono disposizioni specifiche relative alla definizione degli stanziamenti di spesa per i rinnovi contrattuali degli enti del settore pubblico. In aggiunta, il comma 14 dell'articolo 2 prevede che, oltre alle risorse previste dai commi da 9 a 12, le amministrazioni destinatarie utilizzino le risorse disponibili ai sensi dell'articolo 2, commi 33 e 34, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, conseguenti ai risparmi derivanti dai processi di riordino e riorganizzazione delle amministrazioni introdotte dal decreto-legge n. 112 del 2008. Si rileva inoltre che il comma 17 del citato articolo prevede anche che per l'attuazione della sentenza della Corte costituzionale 13 marzo 2009, n. 74, sia istituito un tavolo paritetico tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Regione Friuli-Venezia Giulia e che nell'anno 2010 e per l'importo iscritto nel bilancio dello Stato a legislazione vigente sia corrisposto un acconto di 200 milioni di euro. Infine, l'articolo 2, comma 18, estende agli anni 2010, 2011 e 2012 l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 116, 117 e 118, della legge n. 244 del 2007, laddove si consente alle Camere di commercio di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità ed entro prestabiliti limiti di spesa, determinati in base al proprio indice di equilibrio economico-finanziario, relativi alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. L'articolo 3 reca poi le consuete disposizioni relative alle tabelle da A ad F allegate al disegno di legge e alcune disposizioni di carattere procedurale, aventi rilievo sul piano finanziario e contabile. A tale proposito, in particolare, il comma 7 del citato articolo 3 dispone che le risorse affluite alla contabilità speciale istituita ai sensi del comma 8 dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2009, recante il dispositivo sul cosiddetto scudo fiscale

con particolare riguardo al settore dell'istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi. Sul punto, come rilevato anche dalla Corte dei conti, va rilevato come si prefiguri pertanto un diverso impiego, comunque legittimo, delle risorse che dovrebbero affluire dall'operazione "scudo fiscale" secondo le indicazione fornite dalla legislazione vigente, dal momento che il vigente articolo 13‑*bis* della legge n. 102 del 2009 ne dispone l'integrale destinazione all'attuazione della manovra di bilancio per gli anni 2010 e seguenti. Per quanto concerne invece più specificamente le problematiche inerenti la corretta quantificazione degli oneri, vi invito inevitabilmente alla lettura della nota di lettura del Servizio del bilancio. Sotto il profilo politico debbo altresì aggiungere che i lavori in Commissione, con molti meno emendamenti rispetto agli anni precedenti (nelle finanziarie che conosciamo e che abbiamo conosciuto), hanno lasciato spazio ad un dibattito più aperto sulla sostanza generale della manovra e sui molti aspetti ed effetti economici di ricaduta. Molte anche le inammissibilità, va sottolineato, che infatti hanno portato da circa 800 a circa 550 gli emendamenti stessi. Il punto di equilibrio della discussione che si è svolta in Commissione era e rimane la coniugazione tra rigore e sviluppo: la stabilità dei conti, da un lato, e gli aiuti alle famiglie, alle imprese e in generale alle fasce più deboli, dall'altro. Dunque il patto di stabilità e il debito pubblico, da un lato, con la necessità, dall'altro, di ridurre la pressione fiscale, soprattutto soprattutto alle imprese, per far ripartire l'economia più velocemente, aumentando i consumi e agevolando gli investimenti. Il tema dell'IRAP, ad esempio, è stato uno dei temi centrali nella discussione in Commissione, sia per i numerosi emendamenti presentati da tutti i Gruppi, sia per il dibattito che ne è nato, non solo in Commissione, ma anche sui *media*. Forse quest'ultimo aspetto non è del tutto positivo, perché questa comunque è e rimane la sede nella quale discutere di finanziaria e trarre le conseguenze delle decisioni, soprattutto per le attese del Paese, dalle dalle piccole e medie imprese a Confindustria. La Commissione ha voluto dare un segnale; era logico e corretto che il relatore se ne facesse e se ne faccia portatore in questa sede. Le sfumature, anche di sostanza, fra le varie proposte non sono da poco.

con gradualità diverse tra maggioranza ed opposizione; tale attesa sarebbe mortificata se tutto fosse rinviato alla scadenza dello scudo fiscale. Le strategie, sulle imprese come sulla famiglia, visto che molti emendamenti agganciavano la riduzione dell'IRAP al mantenimento del livello occupazionale, possono essere piccoli segnali e piccoli interventi che, in un periodo - mi si perdoni l'espressione - di vacche magre, danno però il tracciato di un impegno e di una strada da percorrere a medio termine. Oltre all'IRAP, grande spazio hanno avuto il taglio delle tasse sui lavoratori, la scuola, le università, la cedolare sugli affitti (tema peraltro con duplice valenza virtuosa: da un lato, l'emersione del nero e, in proiezione, maggiori entrate); per non dimenticare gli effetti benefici degli accordi che la Guardia di finanza sta raccogliendo in tale ambito con i Comuni del nostro territorio. Poi, ancora, la sicurezza, il dissesto idrogeologico, l'Abruzzo, il patto di stabilità per i piccoli Comuni, l'IVA ridotta sul turismo,

Il Governo ha ragione a sottolinearlo e a preoccuparsene e quindi a fare una finanziaria rigorosa, ma credo che la volontà politica debba tenere conto anche di altri aspetti. Questo è il motivo per cui su tali temi si è inserito anche un blocco di emendamenti apparentemente di «controfinanziaria», ma che non lo sono affatto. Anzi, essi sono organici tra loro, non in contrapposizione al Governo ma aggiuntivi, realizzati dalla maggioranza e, in particolare, dal presidente Baldassarri e da altri senatori, come proposta fattibile ed occasione di sprone e dibattito vero, fatto non di annunci, ma di ipotesi concrete. Si tratta di emendamenti di ulteriore riduzione della spesa pubblica, con la cancellazione dei finanziamenti a fondo perduto per le imprese, dirottando una parte di tutto ciò su innovazione, università, ricerca, occupazione, famiglie ed infrastrutture.

se la sanità nel Paese sia migliorata del 50 per cento. Probabilmente la risposta è no. Da ciò emerge lo spazio per ricavare risorse, nella misura che possiamo ancora decidere nelle prossime ore, ovviamente insieme al Governo, il quale credo abbia preso atto di questa grande disponibilità al dibattito e alla discussione in Parlamento, insieme qualche risposta alle tante, forse troppe, richieste. Seguirò con attenzione la discussione generale e mi auguro che continui il clima generale che credo abbia prodotto in Commissione un discreto lavoro.

Vorrei ringraziare, oltre all'ottima guida del presidente Azzollini, tutta la Commissione per il clima corretto e di reale contributo con il quale ha lavorato presentando

«la recessione mondiale si è arrestata e si sta ora profilando una ripresa, in larga parte grazie al sostegno delle politiche economiche espansive adottate dai principali Paesi». Queste sono le prime parole scritte nel bollettino economico n. 58, l'ultimo, della Banca d'Italia. La ripresa, prosegue la Banca centrale, si prospetta lenta e non immune da rischi. Rimane, infatti, molta incertezza sulla sua solidità. Anche in Italia, lordo nel trimestre estivo è tornato a crescere, dopo cinque trimestri negativi che ne hanno riportato il valore a più di dieci anni fa. però, non si intravede un'inversione di tendenza, né della domanda interna né di quella estera, mentre l'occupazione è attesa contrarsi ancora più fortemente nei prossimi mesi e i conti pubblici conoscono un pesante deterioramento. Questo sintetico giudizio sulla evoluzione della crisi in Italia e nel mondo dovrebbe suggerire a tutti, Governo, maggioranza e opposizione, di non impegnare energie in attività di sterile propaganda per concentrarle, invece, sulle scelte che possono e devono essere compiute ora per accelerare il passo nella fuoriuscita dalla crisi e, soprattutto, per affrontare quei nodi strutturali che da 15 anni rendono difficile il respiro del Paese e, non sciolti, gli impediranno di camminare alla stessa velocità degli altri quando la crisi sarà finalmente superata. A questo scopo, non gioverebbe al Paese e, alla lunga, a mio giudizio, nemmeno alle sorti della stessa opposizione, essere un'opposizione che negasse, o si rifiutasse di vedere, sia i segni di ripresa sia i meriti acquisiti dall'azione del Governo. Anzi, riconoscere gli uni e gli altri per quello che sono, se e quando ci sono, rende più solide e credibili le critiche per la sottovalutazione dei rischi, per le scelte sbagliate o per i mancati interventi. L'ISAE, nel corso della sua audizione, ci ha detto che sono in costante miglioramento gli indicatori di fiducia delle famiglie e, in misura assai più debole, quelli delle stesse imprese. Se la crisi ha provocato un gravissimo deterioramento del sistema delle aspettative (e noi sappiamo quanto nelle economie sia rilevante il sistema delle aspettative), si tratta di una notizia buona,

Il Governo fa bene ad enfatizzare il miglioramento in corso del clima di fiducia, ma fa male - anzi, malissimo - a non utilizzare l'occasione della crisi per approvare, subito, adesso, in questi giorni, la riforma che renda universale il nostro discriminante sistema di ammortizzatori sociali. I dati fornitici nel corso della sua audizione dall'ufficio studi della UIL, elaborati sulle informazioni relative alle cosiddette comunicazioni obbligatorie su assunzioni e licenziamenti, descrivono, signor Presidente, una realtà drammatica. Le imprese hanno ridotto le nuove assunzioni di un terzo nel giugno 2009 rispetto al giugno 2008: si tratta di un terzo di assunzioni Nello stesso periodo, i licenziamenti sono aumentati in un anno del 10 per cento e si concentrano sui contratti temporanei. Le nuove assunzioni sono quasi tutte a scadenza prefissata.

Questa è la tragica realtà del mondo del lavoro in questo momento in Italia e sappiamo tutti che nei prossimi mesi non avremo un miglioramento, perché gli effetti della crisi si manifestano sul prodotto prima che sul terreno della disoccupazione. faremo ora, colleghi della maggioranza, signor Vice Ministro, la riforma per ammortizzatori non discriminatori verso la parte più debole del mondo del lavoro e verso le piccole imprese, allora Il Governo risponde: a crisi terminata. Come se l'avere o meno a disposizione un sistema efficace di protezione per tutti i lavoratori che perdono e non trovano lavoro fosse indifferente, sia al fine di determinare quale Italia può uscire dalla crisi sia per determinare quali siano le potenzialità del Paese in termini di rilancio del proprio sviluppo. Analogamente, è stato ed è da apprezzare l'intervento del Governo italiano - di concerto con quello degli altri principali Paesi - per impedire che il fallimento di Lehman Brothers fosse seguito dal crollo del sistema bancario dell'economia globale: bene le garanzie offerte ai depositanti, bene gli interventi per il rafforzamento patrimoniale delle banche, oberate dagli effetti di leve finanziarie fatte crescere ben al di là di ogni ragionevole prudenza. Male, anzi, malissimo, il rifiuto del Governo di operare - anche utilizzando lo strumento di Cassa depositi e prestiti per una vera svolta nei tempi di pagamento della pubblica amministrazione, la piaga che riguarda il rapporto tra Stato ed imprese nel nostro Paese e che strangola la liquidità delle imprese in una fase nella quale c'è il *credit crunch,* cioè la riduzione della disponibilità di credito. Male il mancato intervento per il rafforzamento dei Confidi e degli strumenti di garanzia sul credito alle imprese. Se il problema è - come è - far ripartire il flusso del credito verso le imprese, queste misure che noi abbiamo proposto e che il Governo e la maggioranza hanno respinto avrebbero potuto già alleviare le condizioni di scarsità del credito in cui versano le nostre imprese. E tanto più potrebbero farlo nel presente e nel futuro prossimo, assai meglio - a proposito di credito - della improbabile Banca del Sud, cui il Governo dedica energie a mio giudizio degne di miglior causa. Se l'opposizione non deve sposare la logica del tanto peggio, tanto meglio - e non mi pare che il confronto di questo anno e mezzo abbia fatto emergere, dalle parti del Partito Democratico, la prevalenza di questo atteggiamento - il Governo e la maggioranza debbono guardarsi dal rischio di sottovalutare la gravità della situazione. Circola, dalle parti del Governo e della maggioranza, una rappresentazione dell'Italia come «Paese che regge meglio di altri» ai colpi della crisi: noi, col nostro manifatturiero, meglio di chi ha un apparato produttivo squilibrato a favore del terziario e dei servizi finanziari in particolare. Noi, con le nostre banche più "provinciali", meglio di chi ha inseguito il miraggio della banca "globale". Noi, che ora soffriamo di più per il crollo del commercio mondiale, ma ripartiremo più forte degli altri con le esportazioni, quando riprenderanno i consumi nell'economia globale. Noi che possiamo giovarci delle enormi manovre espansive di bilancio degli altri Paesi, senza aver peggiorato più di tanto le nostre condizioni di finanza pubblica. Ecco, io vedo il rischio che il Governo si faccia guidare - nel definire le architravi della propria politica economica e di bilancio - da questa rappresentazione della realtà italiana, che mette insieme dati di realtà - è vero che eccelliamo nel manifatturiero; è vero che abbiamo banche solide; è vero che il nostro deficit pubblico è cresciuto nella crisi dell'ultimo anno meno di quello di altri (fatemi dire: ci mancava pure questa)

Alle stesse conclusioni ci conduce l'esame dei dati sulla nostra presenza nel commercio mondiale e di quelli relativi alla misurazione della produttività totale dei fattori. Colleghi di maggioranza, non è una disputa tra chi vede il bicchiere mezzo pieno e chi lo vede mezzo vuoto. La rappresentazione edulcorata della realtà induce il Governo ad assumere l'atteggiamento di chi pensa che in larga misura i problemi si risolveranno da soli, purché si riesca a mantenere sostanzialmente sotto controllo l'evoluzione del deficit e del debito pubblico attraverso una rigorosa disciplina fiscale. Vorrei essere chiaro: noi non critichiamo il Governo perché mantiene disciplina e rigore della politica di bilancio; critichiamo il Governo perché mostra di ritenere che disciplina e rigore debbano derivare da una politica di non intervento, da una sostanziale immobilità. Ecco cos'è la legge finanziaria e la legge di bilancio che avete presentato. Noi invece riteniamo che agli stessi esiti in termini di mantenimento della disciplina e del rigore della politica di bilancio si debba giungere attraverso coraggiose scelte di riduzione della spesa corrente primaria, compensativa di selettivi interventi di riduzione della pressione fiscale sui redditi medio-bassi e sulle imprese e di un aumento - sissignori! - della spesa pubblica in conto capitale, specie per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e per mettere riparo al dissesto idrogeologico. Di fronte al Paese si misurano quindi due linee di politica economica e di bilancio: quella di chi pensa che - date le caratteristiche e le specializzazioni del nostro sistema produttivo e data la rigidità del bilancio non ci siano le condizioni (e, al limite, neppure la necessità, come dice il Ministro dell'economia) di incisivi cambiamenti della politica di bilancio, né dal lato della spesa, né dal lato delle entrate, e quella di chi vuole promuovere questi cambiamenti - come noi - su entrambi i lati, esattamente perché ritiene che riqualificare, rendere più rendere più efficiente e ridurre la spesa sia possibile e necessario al fine di ridurre la pressione fiscale e di realizzare l'infrastrutturazione materiale e immateriale del Paese. Una cosa è certa: se si continua ad operare ai margini delle scelte di bilancio con aggiustamenti sostanzialmente trascurabili, la strada è segnata. Nel decennio 1998-2008 - lo ha ricordato il relatore al bilancio le spese correnti primarie sono aumentate in termini reali, cioè al netto dell'inflazione, del 2,1 per cento all'anno in media. O si è in grado di rovesciare questo andamento o non c'è libertà della politica economica italiana. Non è vero che la piena immobilità è l'unica scelta possibile: quella del cambiamento è altrettanto realistica, specie ora che la crisi ha reso tutti più consapevoli dei rischi incombenti ed ha creato quindi il consenso per scelte che fino a poco tempo fa sembravano impossibili, tanto erano costose politicamente. Se ora, colleghi, nel secondo anno di legislatura, in piena crisi, il Governo sceglie l'immobilità, i tre anni che ci stanno e che vi stanno di fronte saranno tre anni di sostanziale paralisi, perché i margini finanziari e politici per interventi incisivi non si allargheranno allargheranno nel prossimo futuro, ma tenderanno a restringersi. Al contrario, passata la crisi globale, rischiamo di pagare - come sistema Paese - gli effetti di politiche di bilancio e monetarie più restrittive che gli altri Paesi saranno costretti a mettere in atto per cercare di ridurre le le dimensioni della politica espansiva che hanno fatto nel corso di questo anno e mezzo. Questo dunque è il momento e questa - la decisione di bilancio per il 2010-2013 - è la sede. E se l'alternativa è quella tra le due linee di cui si è detto, è del tutto incongruo - per usare un eufemismo - il rinvio delle scelte al momento in cui si conoscerà il gettito dello scudo fiscale. E mi fa piacere che questo concetto sia stato espresso - naturalmente con altre parole - anche dal relatore di maggioranza. Lo devono sapere i colleghi della maggioranza che si sono sforzati di far vivere - a modo loro ovviamente - una linea diversa rispetto a quella di cui il disegno di legge di bilancio e la finanziaria sono espressione: se il riferimento è alle risorse dello scudo, è nella linea dell'immobilità che ci si sta muovendo. Se si vuole la riconversione e la ristrutturazione della spesa, la riduzione della pressione fiscale, allora lo scudo - con le sue entrate *una tantum* - non c'entra assolutamente nulla. Ed è qui al Senato, ora, in prima lettura, che si può decidere il salto di qualità, cioè il mutamento del segno della politica di bilancio del Governo. Se restano così come il Consiglio dei ministri le ha approvate, le leggi di bilancio e finanziaria esprimono una linea rinunciataria, ben rappresentata non tanto dall'entità della manovra netta - un'aggressiva politica di intervento sulla crisi potrebbe e dovrebbe a nostro avviso realizzarsi, nel medio periodo, a saldi di bilancio inalterati quanto dalla completa scomparsa (tecnica e politica) dell'orizzonte triennale delle scelte allocative, che pur aveva costituito, a mio avviso, l'unico effettivo pregio della manovra impostata con il decreto-legge n. 112 del giugno 2008. È come se il Governo ritenesse di non possedere la forza politica e il rapporto con il Paese necessari per governare la crisi, e accettasse di esserne governato. Dal prometeico «ghe pensi mi» come minimo frutto di una certa sopravvalutazione della "potenza" della politica economica di un singolo Stato - alla politica che io chiamo «ambizione zero», quella di cui è espressione questa legge di bilancio e finanziaria. Può così accadere che neppure le scelte di maggiore pregio - operate dal Governo in quest'anno e mezzo o già in vigore al momento del suo insediamento - trovino nel bilancio le risorse adeguate alla loro implementazione. È il caso del definanziamento degli sgravi fiscali sulla quota di salario da contrattazione di secondo livello. È il caso della soppressione delle detrazioni del 55 per cento per gli investimenti delle famiglie in ristrutturazioni edilizie per il risparmio energetico. Tutti diciamo che la modernizzazione delle relazioni sindacali, l'innalzamento della produttività, la soluzione stessa della questione salariale passano per il rafforzamento della contrattazione di secondo livello, che il modello contrattuale del 1993 - cui pure vanno riconosciuti grandi meriti - relega invece in un ruolo subalterno. Tutti ci riempiamo la bocca - destra, sinistra e centro - di *green economy*, la ristrutturazione ecologica dell'economia, del sistema produttivo, del sistema sociale sia per migliorare la qualità ambientale e sociale, sia per dar luogo a nuovi settori produttivi di beni e servizi, ad alta intensità di manodopera e di innovazione tecnologica. E il Governo, alla prima occasione, che fa? Non finanzia né gli sgravi per il salario da contrattazione di secondo livello, né le detrazioni per il risparmio energetico. Non si risponda, per favore: «coi soldi dello scudo, rifinanzieremo», perché questa risposta è la prova provata che si sta seguendo l'approccio della immobilità, dello «zero ambizioni». Crede forse, il Governo, che famiglie, imprese e lavoratori potranno investire soldi, impegno e fiducia in scelte tanto decisive per il loro futuro, se chi dirige il Paese mostra tanta incertezza di orientamento e tanta incapacità di muoversi nell'ottica del medio e del lungo periodo (l'unica che serve di fronte ad una crisi come quella che noi stiamo vivendo)? Anche la recente legge per la riforma della pubblica amministrazione - approvata qui al Senato col contributo determinante delle proposte e delle soluzioni tecniche presentate dal Partito Democratico, così come è accaduto per la legge sul federalismo fiscale - è trattata dal Governo, che pure la esalta astrattamente nella propaganda, con sufficienza: nessuno sforzo per associarvi obiettivi puntuali e verificabili di efficienza e risparmio. Così che tocca al Gruppo del Partito Democratico, come è accaduto e accade in questa finanziaria, presentare emendamenti in sessione di bilancio che fanno leva

della pressione fiscale sulle famiglie e sulle imprese. C'è da chiedersi se Governo e maggioranza si rendano conto che senza intervenire sulla spesa che finanzia la macchina della pubblica amministrazione, il bilancio pubblico italiano, come ha detto il relatore di maggioranza sulla legge di bilancio, non presenta margini per politiche sociali e di promozione dello sviluppo adeguate alle drammatiche urgenze economiche e sociali proposteci dalla crisi. È certamente vero che dalla riforma cosiddetta del federalismo fiscale può venire un robusto contributo a riaprire spazi di libertà

che ha bocciato e ha sciolto la società mista che si era costituita nella Regione Veneto proprio a questo proposito. Ora, nel corso del dibattito

Alla fine, in Commissione, non è stato approvato nulla di effettivamente rilevante. Ma si è sviluppato - partendo da emendamenti spesso molto simili presentati da senatori del Partito Democratico e da senatori del PdL un confronto di merito, non propagandistico, non tra sordi, non inutilmente recriminatorio. Ecco, a fronte di ciò - ne parlerà - a me in questa sede compete una precisazione e una proposta di metodo. Quanto alla precisazione, questa volta nessuno nel Governo può pensare di cavarsela ergendosi a difensore del rigore, contro politiche espansive irresponsabili da attribuire a noi. L'intervento di medio-lungo periodo che ispira le nostre proposte emendative è organizzato attorno ad obiettivi di riduzione della spesa corrente primaria assolutamente realistici e credibili. Né proponiamo di spingerci in pericolose avventure lafferiane, ipotizzando improbabili e mirabolanti effetti di crescita del PIL derivanti da certe ed immediate cadute di gettito. abbiamo proposto - per la riduzione della pressione fiscale - soluzioni che intanto la realizzano (penso all'IRAP), in quanto se ne siano create le condizioni finanziarie, attraverso proporzionali risparmi. che ha il grande pregio di piazzare davanti alla porta del Governo - quale che esso sia - ogni giorno di ogni anno i portatori di legittimi interessi economici che pretendono il conseguimento di quegli obiettivi di risparmio cui sono associati i loro sgravi fiscali. alla proposta di metodo, e la ringrazio, signor Presidente, per i minuti che mi ha concesso in più. Se il Presidente del Consiglio - come ha non detto, ma scritto nel suo messaggio all'assemblea della CNA intende introdurre una significativa correzione alla sua politica economica e di bilancio, lo faccia in modo trasparente adesso, prima promuovendo il confronto interno alla sua maggioranza, poi portandone gli esiti in Parlamento, durante la sessione di bilancio. Noi, per parte nostra, in modo altrettanto trasparente, parteciperemo al successivo confronto, senza forzature e senza strumentalizzazioni. Se invece la maggioranza cercherà di agire senza chiarezza e senza trasparenza magari con un bell'ordine del giorno finale che, qui al Senato, rinvia al momento magico delle entrate derivanti dallo scudo fiscale ogni soluzione ed ogni scelta, compresa quella sul carattere di fondo della politica di bilancio, che con lo scudo non c'entra nulla - sarà l'intero Paese a perdere un'altra importante occasione.

già consegnato una relazione scritta e dopo l'intervento del senatore Morando, mi limiterò solo ad alcune considerazioni, in modo da recuperare anche parte del tempo. Il relatore di maggioranza parlava di una finanziaria snella: il termine più appropriato sarebbe anoressica, perché in questa finanziaria in realtà non c'è nulla:

considerazioni di tipo diverso. I vari Stati hanno anche agito in maniera differente: c'è chi ha atteso e chi, invece, ha fatto politiche attive per affrontare la crisi. Abbiamo dunque uno scenario diversificato, così come diversi sono anche i giudizi.

una discussione. Penso che noi dobbiamo dimostrare che stiamo padroneggiando la situazione e che siamo consapevoli della profondità della crisi. La fiducia agli italiani la diamo non tanto se lanciamo messaggi di ottimismo, ma se facciamo vedere come classe politica che abbiamo ben presente quali sono i problemi del Paese e che

quindi se vogliamo porci questo problema e, attraverso una politica seria di detrazioni, riuscire a ridare un po' di potere d'acquisto ai redditi e alle pensioni più basse,

potervi fare fronte con lo scudo fiscale? Insomma, se vogliamo prenderci in giro, possiamo farlo, ma non è questo il modo di affrontare la situazione!

questo Paese ha infatti nel turismo e nell'agricoltura due valori aggiunti che sono importantissimi e fanno girare l'economia. Il turismo è

*(PD)*. Signor Presidente, onorevole vice ministro Vegas, colleghi relatori e senatori, Schumpeter, all'inizio del Novecento, affermava che il bilancio dello Stato è lo specchio di tutti i problemi politici e sociali di una Nazione. È attraverso le tabelle poco attraenti del bilancio che si esplica la politica economica che lo Stato persegue; dal bilancio ricaviamo quali sono le politiche di stabilizzazione, di crescita, di redistribuzione e riallocazione delle risorse. E cosa ricaviamo, signor rappresentante del Governo e signori della maggioranza, da questo bilancio dello Stato e dalla legge finanziaria del 2010? L'intervento proposto dal Governo, a fronte della più profonda recessione dal dopo guerra ad oggi, è stato fondamentalmente nullo. Eppure, anche a voi dovrebbe essere noto che il 2009 è stato l'anno più duro della storia economica italiana dell'ultimo secolo: il PIL ha subito una caduta del 4,8 per cento, il rapporto fra *deficit* e PIL

in più in un solo anno e senza alcuna manovra di sostegno all'economia!). In tema di lavoro, i ricorsi alla cassa integrazione ordinaria sono al 300 per nel periodo da gennaio a settembre 2009, le imprese hanno ridotto le nuove assunzioni di un terzo, i licenziamenti sono aumentati del 10 per cento, le nuove assunzioni sono quasi tutte a scadenza prefissata (ben 4 nuovi rapporti di lavoro su 5 sono a tempo determinato), per cento dei contratti del precariato sono trasformati a tempo indeterminato. In questo contesto le leggi finanziaria e di bilancio non hanno previsto alcuna misura di sostegno all'economia. La finanziaria "snella", in realtà,

Come affermato dal nostro relatore di minoranza, noi non critichiamo il Governo quando mantiene disciplina e rigore nella politica di bilancio, ma quando afferma che i problemi si risolveranno da soli, sol che si mantengano disciplina e rigore. Critichiamo il Governo perché ha optato invece per una politica economica di non intervento e di immobilità di fronte alla più grave recessione mai verificatasi dal dopoguerra ad oggi. Nulla, signori della maggioranza, avete previsto per il sostegno all'economia reale: tutto è rimandato ai saldi che deriveranno dalle entrate dello scudo fiscale, che però - come ci insegnate - è una misura *una* *tantum*, sulla quale non è possibile fondare una sana politica economica e di bilancio. con il collega Legnini e altri autorevoli senatori del mio Gruppo, ho presentato 16 emendamenti per rendere la ricostruzione post‑terremoto in Abruzzo certa ed estesa a tutti gli aventi diritto: ebbene, ne avete ammessi sette.

per gli sfollati, peraltro ad oggi ancora insufficienti e che rischiano di diventare l'unica e definitiva soluzione alloggiativa per le popolazioni terremotate. Il decreto-legge n. 39 del 2009 ha rappresentato una risposta parziale, affatto esaustiva alla futura ricostruzione: troppe le fattispecie non contemplate dal decreto convertito, numerose e di sostanza le differenze tra il sistema di norme e garanzie poste in essere nel confronto poste in essere nel confronto fra la ricostruzione in Abruzzo e quella realizzata in Umbria e Marche per il terremoto del 1997. La motivazione che ispira le nostre proposte non è quella di venire meno alle politiche del rigore, né quella di "assalire la diligenza", bensì di pensare ad un modello di organizzazione della ricostruzione con l'equità, la solidarietà e la maggior efficienza ed efficacia possibili, quali sono richieste in un dramma simile. una ricostruzione che non lasci l'Abruzzo, e la provincia dell'Aquila in particolare, impoveriti da una calamità non richiesta, ma lo instradi su un sentiero di rinascita, verso una crescita sostenibile. Infatti, se è drammatica la situazione dell'economia italiana, ancor più lo è quella della Regione Abruzzo, colpita dalla crisi internazionale, dalla caduta dell'*export* e dagli effetti devastanti del terremoto.

conoscere con quali fondi verrà sostenuta la ricostruzione delle case di abitazione o delle case degli emigrati non residenti, dei luoghi di lavoro, degli esercizi commerciali, degli studi professionali e delle piccole e medie imprese, insomma,

Per il terremoto di Umbria e Marche del 1997, signor Presidente, la sospensione del pagamento è durata 12 anni, non otto mesi e il recupero chiesto ai terremotati di quelle Regioni, iniziato solo il 1° luglio 2009, fu pari al 40 per cento degli arretrati; in Abruzzo, signor presidente Schifani, la sospensione del pagamento dei tributi è fissata in otto mesi, con il recupero del 100 per cento degli arretrati a partire dal 1º gennaio 2010 e in sole 24 rate. Lo scorso luglio, durante i lavori parlamentari per la conversione in legge del decreto-legge n. 78, non avete dato parere favorevole nemmeno ad un ordine del giorno sulla restituzione delle imposte, con il quale vi sareste dovuti impegnare a modificare l'articolo 8-*bis* di quel decreto, in sede di un prossimo decreto‑legge emanando: ci proponeste di scrivere non «nel prossimo», ma «in uno successivo». Ad oggi, avete emanato altri quattro decreti-legge e non avete la minima intenzione di modificare questa vergognosa norma a danno dei terremotati abruzzesi, con la quale - glielo ricordo, signor vice ministro Vegas - finanziate la ricostruzione: quella che non avete finanziato nel decreto-legge, volete finanziarla con le entrate e con la restituzione delle imposte! Ripensate al parere e al voto sull'emendamento 2.185 e sottoscrivetelo, colleghi della maggioranza, fatelo diventare patrimonio di tutto il Senato, e non di una parte soltanto di quest'Aula. Riportate i tempi di sospensione e restituzione dei tributi per le popolazioni del cratere sismico e per quelle che hanno subito danni diretti o indiretti causa del sisma, così come è stato fatto per Umbria e Marche, al fine di favorire la ripresa dell'economia reale per quei territori. La drammatica situazione economica impone di passare subito ad un'economia del terremoto, possibile solo se le imprese locali riusciranno a svolgere quel ruolo chiave che loro compete nella filiera produttiva. In questo senso, il finanziamento delle zone franche urbane con l'emendamento 2.234, da voi respinto in Commissione, serve soltanto a risolvere questo problema. L'economia della terremotata provincia de L'Aquila è oggi ad un bivio. Con le zone franche urbane potrà migliorare il futuro delle piccole e medie imprese, dei commercianti, degli artigiani e dei professionisti, solo se le risorse assegnate dal Governo saranno aumentate. Tutti ve ne saranno grati, non una sola parte politica. Se ciò non accadrà, L'Aquila e i Comuni colpiti dal terremoto diventeranno territori morti e con essi i Comuni contigui, senza alcuna possibilità di ripartire. Avete respinto, infine, l'emendamento 2.391 sulla tratta ferroviaria Pescara-Roma. Era già legge dello Stato, signor Vice Ministro; l'avete cancellata per finanziare il primo decreto-legge del Governo Berlusconi. A torto o a ragione, ci proponete ancora un ordine del giorno, che vi impegna formalmente e non vi obbliga a fare nulla. Ditelo ai cittadini abruzzesi, italiani anch'essi, che non arrivano in tempo al lavoro o all'università per i ritardi e le soppressioni in misura ben superiore alla statistica, che non entrano in autobus o in auto a Roma, perché dal congestionato casello di Roma Est non si entra nel territorio urbano di Roma, che spopolano i piccoli Comuni per andare ad ingolfare, con le giovani coppie, la periferia romana. Ditelo a loro, ditelo a questi cittadini che la risposta della maggioranza che sostiene il Governo Berlusconi, con questa legge finanziaria per il 2010, per far ripartire l'economia abruzzese dalla pesante crisi economica e dal terremoto, si chiama ordine del giorno!

Signor Presidente, colleghi, come evidenziato dal mio Gruppo in più occasioni nel corso di questo lungo periodo di crisi e nello stesso dibattito che accompagna l'esame dei presenti provvedimenti finanziari, l'attuale politica del Governo sul fronte del contenimento della spesa, senza i necessari interventi di natura strutturale, in grado cioè di affrontare una crisi che non ha certo natura congiunturale, determina - come abbiamo visto - un abbassamento del tasso di crescita e un progressivo aumento del debito. Accanto a misure di natura strutturale su questo fronte, esiste poi, come abbiamo sottolineato con insistenza, la necessità di garantire al Paese - dentro la crisi - la coesione sociale, poiché è altissimo il rischio di una sua ulteriore frammentazione, di una ancora più marcata divisione fra le aree della penisola e fra le varie categorie sociali, a cominciare da chi meno ha, da chi si trova in condizioni di lavoro precario, da chi è in cassa integrazione o è disoccupato. Da qui l'esigenza di misure che riescano non solo ad intervenire in modo strutturale sul fronte della spesa pubblica, ma che, a partire dai redditi medio-bassi e dalle famiglie, possano aiutare la stessa ripresa del ciclo economico e la crescita. A tale proposito voglio ricordare, signor Presidente, la grande manifestazione svoltasi a Roma nei giorni scorsi, promossa da tutti i sindacati della Polizia di Stato e del Corpo forestale, cui hanno espresso la loro solidarietà anche le rappresentanze elettive del personale militare. In quella iniziativa si è alzata forte la voce contro la politica del Governo, che con i tagli indiscriminati al settore sta portando al collasso tutto il comparto della difesa e della sicurezza, e si è espressa altresì una preoccupazione per la mancanza di risorse per i rinnovi contrattuali. Ricordo che una larga percentuale dei 550.000 operatori del comparto sicurezza e difesa è inquadrata nei parametri iniziali del ruolo delle truppe (per le Forze armate) e in quello degli agenti (per le Forze di polizia), con stipendi medio-bassi, dai 1.200 ai 1.600 euro netti al mese. Non rinnovare i contratti significa deprimere ulteriormente il tenore in vita di questi operatori e delle loro famiglie e, sul piano economico, ridimensionarne ulteriormente i consumi. Venendo allo specifico del comparto Difesa, la manovra prevede la conferma di pesanti tagli all'esercizio e al reclutamento, scarsissime risorse per i rinnovi contrattuali e un'assenza totale di interventi nell'area industriale della Difesa. Il tutto senza una vera e propria strategia di riqualificazione e razionalizzazione della spesa per il comparto. Il Governo si dimostra, ancora una volta, non in grado di intervenire sulla qualità e sulla composizione della spesa militare, così da arrestare l'evidente decadimento operativo dello strumento militare, ammesso dalla stessa maggioranza. Anche in questa occasione, mancano volontà e capacità di produrre quelle necessarie innovazioni, anche di natura strutturale, che possano fare di questo settore primario del nostro Paese un luogo utile non solo a garantire difesa e sicurezza, ma anche sviluppo e crescita qualitativa della nostra stessa economia e, più complessivamente, della nostra società. Per quanto riguarda il comparto Difesa, siamo quindi di fronte ad una situazione paradossale. Il Governo ha di fatto trasformato, attraverso i tagli di bilancio, il nostro strumento militare, che il Parlamento aveva definito con un assetto organico pari a 190.000 militari. Oggi è giunta notizia che il presidente della Repubblica Napolitano ha convocato per l'11 novembre il Consiglio supremo di difesa, per la presentazione dei risultati della Commissione di alta consulenza e studio per la ridefinizione complessiva del sistema di difesa e sicurezza nazionale. Vedremo in quella sede finalmente qual è la linea politica del Governo per il comparto Difesa, quale modello viene proposto. Nel frattempo, però, in assenza di qualunque elaborazione e di una vera politica di difesa, l'attuale modello è stato già modificato con il taglio degli organici e delle risorse per il reclutamento e l'esercizio, e portato, come si legge negli stessi documenti governativi che accompagnano la manovra, sull'orlo dell'ingovernabilità. Con tutta evidenza, ciò contrasta con il ruolo che nella vita pubblica interna e nella politica estera, nelle missioni internazionali, come ha ricordato il presidente Napolitano oggi, nella ricorrenza del 4 novembre.

ben 4-5.000 soldati, già in servizio da diversi anni, potrebbero essere licenziati, ignorando la loro legittima aspettativa di transitare nel servizio permanente delle Forze armate o nelle forze di Polizia. Si tratta, signor Presidente, di personale, composto interamente da giovani trattenuti in servizio, che ha svolto il compito assegnato con professionalità e sacrificio, spesso a rischio della vita stessa. Ancora, ma non da ultimo, con un *blitz* notturno, a quanto pare nemmeno concordato all'interno della stessa maggioranza, è stato inserito nella finanziaria un emendamento con cui si costituisce la società Difesa servizi Spa. Difesa servizi Spa. Essa ha un vizio di fondo, che trae origine dalla storia stessa di questa norma, presentata due volte sotto forma di emendamento, poi come disegno di legge, cui è stata abbinata una nostra proposta alternativa, e ora presentata di nuovo come emendamento alla finanziaria. In sostanza, si è sempre tentato di eludere il confronto parlamentare di merito, espropriando la Commissione difesa delle proprie competenze. Si tratta di un nuovo soggetto, una società per azioni, destinata a gestire l'acquisizione di beni e servizi per la Difesa e le altre Forze di polizia, e a rivestire il ruolo di centrale di committenza per tutto il comparto. Sul piano formale, si rileva che detto emendamento è stato inserito con una forzatura delle norme di contabilità pubblica volute dallo stesso centrodestra. Allo stesso tempo, tale emendamento introduce in modo del tutto discutibile una norma a carattere ordinamentale che, senza alcun approfondimento, modifica sostanzialmente il ruolo pubblico della Difesa, sottraendo alcune precise prerogative agli attuali organi competenti. Inoltre, sempre per quanto riguarda la forma, sono sette mesi, signor Presidente, che in Commissione difesa si lavora su questo tema: stati depositati due disegni di legge e si sono svolte decine di audizioni. Si è voluto quindi eludere o fuggire dal confronto parlamentare, ricorrendo a questo espediente. Nel merito della norma in questione, si sottolinea il fatto che la funzione precipua di questa società per azioni è quella di fungere da canale di esternalizzazione di lavori e servizi. Risorse pari a circa 3 miliardi e mezzo di euro all'anno vengono consegnate a tale società per azioni, che potrà agire in regime privatistico, evitando ogni controllo, con evidente rischio per la trasparenza e la correttezza dell'azione amministrativa pubblica. Si evidenzia, ancora, che lo statuto della società potrà essere modificato senza alcun controllo parlamentare. Il fatto che una simile importante operazione venga effettuata con un emendamento alla finanziaria, in assenza di relazione tecnica, solleva molti e gravissimi dubbi, con riferimento al perimetro dei compiti della società stessa e all'impatto della sua operatività per il bilancio dello Stato. Signor Presidente, mi permetto di segnalare all'attenzione dell'Aula che dalla finanziaria 2004 questa è la prima volta che non trova riscontro nei documenti di bilancio la copertura del fondo di riserva per le missioni internazionali. Per il prossimo anno, quindi, la proroga delle singole missioni internazionali di pace dipenderà interamente dalle autorizzazioni di spesa del Ministro dell'economia e delle finanze che dovrà, di volta in volta, trovare la necessaria copertura finanziaria.

il mio contributo al dibattito verte sulla spesa di un importante settore. Tra l'altro, in questi giorni ci siamo resi conto che l'argomento principale e preponderante trasferito nel dibattito del Paese in questa congiuntura è esattamente la riduzione della spesa. Il parere della Commissione igiene e sanità sui disegni di legge di bilancio e finanziaria per il 2010 si è sviluppato, il 13 ottobre scorso, in una visione definita scoraggiante dalle opposizioni, a causa della rottura verificatasi tra Governo e Regioni sul Patto per la salute. Indubbiamente, si proponevano riflessioni circa colpe ascritte al Governo in quanto insensibile, per una immaginaria riduzione di risorse e per un antifederalismo pratico, in quanto esso decideva tagli a propria discrezione, senza consultazione con le Regioni, dimentico di salvaguardare il futuro del servizio pubblico sanitario. Un'accusa chiara di interesse a sviluppare il privato contro il pubblico. Pur contestando queste affermazioni, esagerate nella preoccupazione e - spero involontariamente - portate ad indurre insicurezza nella tutela della salute dei cittadini, soffrivo nel confronto per il fatto che, a quella data, il Patto per la salute non era ancora stato firmato. Il tavolo delle trattative era stato bruscamente interrotto. Oggi, dopo il 23 ottobre, a "patti" firmati, posso confermare la comune sensibilità nella Conferenza Stato-Regioni, esaltata anche nell'azione del Governo, che con le Regioni conferma non solo la quota finanziaria del 6,37 per cento del PIL, ma trova le opportune integrazioni con i suoi impegni formali oltre il dato secco già stabilito nella finanziaria 2007, pur iscrivendo l'accordo e le risorse di questo disegno di legge in una cornice economico-finanziaria che risente, ovviamente, della crisi internazionale. L'attuale Patto per la salute a ridosso della legge finanziaria pone la cornice ideale nella quale si introducono meccanismi più idonei nelle modalità di gestione della spesa sanitaria. Non si possono pretendere in questa sede regolamentazioni e programmazioni. La dotazione per detta spesa è stata ritenuta, in molti contesti, più che congrua anche da autorevoli esponenti dell'opposizione, ma condivido con loro la necessità di valutare senza pervenire ad una riforma organica del Servizio sanitario nazionale, anche in considerazione del fatto che non sono mature al momento adeguate condizioni economiche e culturali - l'avvio - l'avvio di processi di riorganizzazione, d'intesa con le Regioni, per riqualificare progettualmente la spesa. Più che incrementare il Fondo, bisogna spendere meglio con maggiore responsabilizzazione e non vanno disgiunti interventi sanzionatori per chi si allontani da questo principio, rivedendo l'attenzione nei commissariamenti, che nel "Patto" si confermano, e nelle sanzioni con cui le popolazioni di vecchie e nuove "Regioni canaglia" si verranno a trovare loro malgrado. Negli accordi, vi è non solo la riduzione di posti letto - misura talvolta adottata in passato in modo indiscriminato, senza valutare i dati ambientali e d'uso, determinando carenze e sofferenze - ma, come ben suggerito da Governo e Regioni, si fa riferimento a *standard* di strutture regionali e nazionali. Questa è la riduzione proposta. Non è secondario il richiamo a rivisitare le politiche per il personale. non sono solo carenze numeriche, rilevanti negli effetti di efficienza ed efficacia del Servizio sanitario nazionale, anche per rispettare i principi della Suprema Corte,che a questo ci richiama, in riferimento alla tutela della salute del paziente attraverso prestazioni d'opera di personale con giuste

essendo efficace questo Servizio nazionale, ma rispetto a questo, signor Vice ministro, anche con le finanziarie, anche con il Patto della salute, bisogna creare i momenti di vigilanza, pur ribadendo che non è una spesa da aumentare. Bisogna spendere però in modo più giusto, più adeguato, più controllato, più incisivo, più opportuno. È altresì opportuno, come emerso tra l'altro nel dibattito in Commissione igiene e sanità, che a questo fine si chieda al Governo di rivedere anche i sistemi di selezione di ammissione alla facoltà di medicina e chirurgia, in modo più appropriato alle finalità di selezione numerica

nel controllo degli accessi devono essere riaperte guardando al numero ed alla qualità. Si rivedano, altresì per i laureati i percorsi di accesso alle specialità, coprendo settori ormai deficitari da tempo (come anestesia, radiologia, cardiologia ed altre branche) e si provveda, soprattutto per le branche chirurgiche, a realizzare norme che garantiscano *tutor* e specializzandi nella graduale assunzione di responsabilità. Dopo 11 anni di studi universitari, frequentemente immettiamo medici, personale sanitario che dovrebbe esser in grado di intervenire, ma che necessita di altri 10 anni per formarsi in modo adeguato. Qualcosa non va, e ce ne siamo accorti nei rapporti con l'Europa, soprattutto negli ultimi tempi. Dal prossimo anno nelle nostre università, nei nostri percorsi

l'istituendo Dicastero della salute dovrà rendersi interprete di queste necessità nell'uso delle risorse in collaborazione con il MIUR, controllando anche a tal fine il giusto uso delle finanze, per spendere meglio le risorse che ci sono e che sono preziose. È certamente importante, senza volere ripetere che non è maturo il tempo per una riforma globale, che la medicina territoriale riprenda vigore nella traduzione delle norme finanziarie, finalizzate a pratiche di salute concrete extraospedaliere. Occorre forse un intervento di controllo e vigilanza dello Stato proprio per tutelare meccanismi ormai riconosciuti in ogni dove, di primaria risposta ai bisogni di salute attraverso interventi territoriali. Tutto ciò nelle conferme date anche nel "Patto per la salute" che riapre, tra l'altro, l'importante capitolo della programmazione edilizia sull'ex articolo 20 della legge n. 67 del 1988. Mai più - signor Vice Ministro - interventi a pioggia per politiche di campanile, senza risposte ai bisogni reali con l'articolo 20. Ci fu una grande ripresa, almeno al Sud, dei lavori pubblici attraverso questo articolo, ma non sempre vi è stata corrispondenza con una migliore logistica e funzionalità sanitaria. Le emigrazioni sono continuate talvolta anche per le sole condizioni alberghiere. Non si è partiti dal Sud per grandi interventi al Nord. Talvolta si è partiti anche per un banale intervento di appendicectomia perché perché le condizioni erano molto più dignitose per poter tenere casomai il bambino e la madre in quell'ambiente. L'ex articolo 20 - oggi che si riparte

Si dovrà intervenire su questi ospedali in modo prioritario. Quello dell'articolo 20 sia un intervento globale e coordinato. Si vigili affinché questi interventi siano finalizzati ad azioni fondamentali ed alla prevenzione di disastri, rispetto ai quali spesso si interviene solo successivamente. Poco si fa, infatti, per prevenire e consolidare un soccorso sicuro nel momento delle Occorre che queste risorse, rimaste importanti, siano controllate nella spesa proprio per produrre risultati corrispondenti ai soldi pubblici che si impegnano. Bisogna superare il luogo comune per cui in sanità ormai si trova l'unica zona franca per la corruzione incontrollabile e silenziosamente

il relatore Latronico nella relazione al bilancio diceva che, dato il contesto di incertezza, il Governo ha scelto una linea di forte prudenza per evitare gli effetti indesiderati di manovre espansive; ne deriva, a seguire e conformemente, il profilo della legge finanziaria. Dunque, direi che il nostro rischia di essere un dibattito parlamentare sul nulla. Nulla di fatto per quanto riguarda la consistenza della manovra, ma nulla nel senso di vuoto anche per quanto riguarda la prospettiva: un'idea di Paese, un'idea di futuro almeno prossimo per l'Italia. Questa è la cosa più grave e la responsabilità più pesante del Governo in questo triste autunno italiano, che preannuncia un inverno ancor più triste e freddo per tante famiglie, non solo meridionali e non solo terremotate. Nei pochi minuti che ho a disposizione non voglio insistere tanto sulle nostre proposte, che sono serie e sono state chiaramente presentate dai relatori di minoranza, proposte che configurano un'altra finanziaria possibile e sostenibile, una finanziaria capace di supportare il lavoro, le famiglie, le imprese, i redditi in questa lunga e difficile crisi. Mi limito a dire che fin dall'inizio della crisi, che ha coinciso con l'avvio di questa legislatura, il Governo si è distinto per non aver mai voluto prendere in considerazione, non dico la nostra proposta complessiva, ma nemmeno una delle nostre proposte, anche solo per discuterla e verificarne la praticabilità. Anche in questa occasione in Commissione bilancio (mi auguro fin d'ora che, come è stato detto anche dal relatore Saia, le cose possano cambiare nel dibattito al Senato) il Governo ha risposto con un *niet* a tutte le proposte dell'opposizione e su tutta la linea; questo rapporto predicato e agito dal Governo nei confronti dell'opposizione non è certo un buon indicatore per lo stato della nostra vita democratica. La vita democratica, la qualità e la produttività del lavoro nelle istituzioni, il clima istituzionale non è completamente altro dal Paese reale. La nostra Italia negli ultimi trent'anni non è mai stata tanto divisa e tanto diseguale, spesso avvilita e spesso incattivita, come ora. Come non vederlo? È una realtà che tutti possiamo toccare con mano. E come non vedere che gli inviti all'ottimismo, gli appelli alla fiducia del Presidente del Consiglio e le manovre economiche all'insegna dell'aspetta e stai a vedere, immaginando magari di poter ricavare qualche beneficio indiretto dalle politiche espansive degli altri Paesi europei, sono tutte franate, tanto erano evidentemente fondate sul nulla. E mentre ancora una volta la maggioranza cerca di indorare la pillola con la propaganda di una rapida e certa fuoriuscita dalla crisi nel 2010, il Paese reale i conti con la crisi li fa sul serio e sa che non sarà facile risalire la china. Quando penso al Paese reale penso al territorio in cui vivo, Napoli, la Campania, che a qualcuno fa evidentemente tanto comodo descrivere unicamente ed esclusivamente come l'impero del male, dell'immoralità

penso a Castellammare di Stabia senza Fincantieri, e a tante altre aziende importantissime nella provincia di Napoli, come Montefibre, Eutelia, Unilever: l'elenco è lunghissimo. Quante decine di migliaia di famiglie coinvolte, famiglie dove il reddito è spesso solo quello del capofamiglia; e quante comunità sconvolte, territori desertificati che diventerebbero campo libero esclusivamente per l'azione criminale. Sono 15.700 i cassaintegrati in deroga nella mia Regione e in un anno sono stati perduti 108.000 posti di lavoro. Penso ai lavoratori socialmente utili, perché nella legge finanziaria non vengono rifinanziate le leggi che li sostenevano e questo vuol dire che migliaia di persone resteranno Penso anche al disastro della scuola pubblica con gli 8 miliardi di euro tagliati in tre anni a livello nazionale, con 132.000 posti di lavoro in meno, moltissimi nella mia Regione. A questo proposito io capisco tutte le difficoltà incontrate dal ministro Gelmini e se dipendesse da lei probabilmente non avrebbe inferto alla scuola il più grande licenziamento di massa della storia storia della Repubblica, ma quando la sento parlare mi chiedo perché continua con la litania che la scuola non sarebbe un ammortizzatore sociale: una litania che suona come un'offesa per tanti insegnanti che hanno dato tantissimo alla scuola italiana, restando precari per anni e oggi definitivamente esclusi dalla scuola stessa. Anche così, umiliando le persone, cresce la sfiducia; sfiducia che, come fenomeno sociale, aggrava certamente la crisi in atto. Il Partito Democratico in quest'Aula è stato profeta inascoltato con le sue proposte e con l'idea, che riproponiamo anche oggi, di non perdere l'occasione che la crisi ci offre di sviluppare la coesione tra noi, di spingere ad unirci e costruire politiche tali da innestare una crescita più dinamica, una prospettiva di risanamento, scambiandola anche con la previsione di un aumento di deficit e di debito transitorio nonché del suo rientro certo e programmato.

il rapporto stretto tra il debito e la bassa potenzialità di crescita. Come si esce da questa stretta tanto grave? La proposta di cui si sta discutendo in queste ore, secondo i giornali, e cioè un minitaglio dell'IRAP, attualmente allo studio insieme a qualche altra misura debolmente finanziata, evidentemente sono ben poca cosa, ma quello che davvero manca è una visione e anche una *leadership* capace di unire il Paese in uno sforzo comune all'altezza dei problemi gravissimi che abbiamo di fronte. La crisi non è un incidente di percorso. Molti nel mondo e in Italia la raccontano come come una crisi esclusivamente finanziaria e di un modello che certo va corretto ma non va modificato. Quello che non si vuol vedere è che non regge più un modello economico dove il prezzo della crescita è l'aumento progressivo delle diseguaglianze e delle differenze di reddito tra ricchi sempre più ricchi e poveri sempre più poveri. Paese, dove le diseguaglianze erano diminuite fino al 1982, oggi è ai primi posti in Europa per l'aumento delle diseguaglianze, la concentrazione della ricchezza e il divario fra ricchi e poveri. La lotta alle diseguaglianze crescenti, la riduzione del divario tra grande ricchezza e grande povertà è un fattore decisivo di coesione sociale, è un tema al quale riconduce anche la nostra Costituzione e rispetto al quale verificare gli impatti delle nostre azioni per la crescita economica. Superare le barriere ideologiche del passato e porre questo tema non a sinistra ma al centro della politica e dell'azione di governo è l'impresa da compiere per la formazione di una nuova classe dirigente all'altezza dei tempi, delle attese e dei bisogni di oggi. n. 533, nonché del parere della Giunta per il Regolamento espresso nella seduta del 7 giugno 2006, all'attribuzione del seggio resosi vacante nella Regione Umbria, a seguito delle dimissioni del senatore Leopoldo Di Girolamo, ha riscontrato, nella seduta odierna, che il candidato che segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo della lista a cui apparteneva il predetto senatore è: per la Regione

*(IdV)*. Signor Presidente, colleghi, vice ministro Vegas, la mia analisi dell'impatto dei presenti provvedimenti sul mondo del lavoro sarà purtroppo alquanto semplice. Non si ritrova infatti, nei provvedimenti che oggi siamo chiamati a discutere dopo il primo passaggio parlamentare presso le Commissioni del Senato, nessuna novità significativa rispetto al momento della loro approvazione da parte del Consiglio dei ministri. Non un accenno ad una politica seria per affrontare la crisi, tutt'altro che superata; non un accenno a soluzioni per i gravi problemi del mondo del lavoro. Al contrario, possiamo rilevare come gli interventi più significativi in merito sono costituiti da un taglio drastico delle risorse per alcune importanti voci di bilancio (come il Fondo per l'occupazione) e il rinvio - di fatto *sine die* - del rinnovo dei contratti del comparto pubblico. Mi scuseranno dunque i colleghi che già conoscono e condividono le nostre posizioni, se saremo costretti a ripetere ancora una volta considerazioni già più volte espresse. Proprio in quest'Aula, poco meno di un mese fa, in discussione sulla Nota di aggiornamento al DPEF per gli anni 2010-2013, avevamo lanciato un allarme, un allarme, basato non su impressioni o visioni ideologiche, ma sulla semplice lettura delle cifre che fotografavano e tuttora fotografano una drammatica realtà. Avevamo riportato i dati e le previsioni del Fondo monetario: disoccupazione

Avevamo riportato la denuncia dello stesso Fondo monetario del pericolo di una *jobless recovery*, cioè di una ripresa senza occupazione. Avevamo ricordato come a livello nazionale i dati e le previsioni dei maggiori istituti preposti al monitoraggio del mondo del lavoro (ISTAT, INPS, CNEL) fossero sostanzialmente concordi nell'indicare nella spaventosa cifra di 500.000 unità il numero dei disoccupati in Italia per la fine del 2009;

e l'avvicinarsi della scadenza delle 52 settimane di cassa integrazione ordinaria per centinaia di migliaia di lavoratori. Qualche giorno fa l'ISTAT ha pubblicato i dati su «Lavoro e retribuzioni nelle grandi imprese» relativi al mese di agosto 2009. Ancora una volta tali dati confermano la tendenza negativa in atto. Infatti, a fronte di un incremento minimo delle retribuzioni, si deve registrare un significativo calo dell'occupazione e delle ore effettivamente lavorate per ciascun dipendente, accompagnate da un incremento delle ore di cassa integrazione ordinaria e di un aumento, seppur minimo, del costo del lavoro. Particolarmente grave si conferma la situazione per quanto riguarda il settore delle grandi imprese dell'industria, dove nei primi otto mesi del 2009 si registra un vero e proprio crollo dell'occupazione. Il Governo e la maggioranza tuttavia, anziché affrontare le questioni appena segnalate, hanno sprecato un intero mese in sterili polemiche interne (tra cui quella a nostro giudizio più vergognosa rimane quella innescata dalle strumentali dichiarazioni del ministro Tremonti sul posto fisso) e in miopi tatticismi, tutti volti alla mera definizione delle future geometrie elettorali in vista del voto amministrativo di primavera. Veniamo ora al merito dei provvedimenti in esame, iniziando dal bilancio dello Stato. Anzitutto vogliamo riproporre in questa sede una questione già da noi sollevata durante l'esame del provvedimento in 11a Commissione e e sulla quale il Governo non ha dato ancora spiegazioni esaurienti. Nell'ambito del programma 1.3 «Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione ed al reddito» mi riferisco al capitolo di bilancio 7206, recante il Fondo per l'occupazione - viene operata una variazione negativa in termini di competenza, rispetto alle previsioni assestate per il 2009, di circa 707 milioni ed una variazione negativa in termini di cassa, rispetto alle previsioni assestate per il 2009, di ben 1.424 milioni.

del decreto legge del 29 novembre 2008, n. 185, le risorse del Fondo per l'occupazione affluiscono al Fondo sociale per occupazione e formazione, che è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro.

Tuttavia, nel provvedimento che stiamo esaminando, il capitolo di bilancio recante il Fondo sociale per occupazione e formazione non c'è. Ribadiamo, come già fatto in Commissione, la nostra richiesta di spiegazioni al Governo. anzitutto perché non sia stata data evidenza contabile al Fondo sociale per occupazione e formazione; in secondo luogo dove siano confluiti gli oltre 700 milioni sottratti dal capitolo 7206 recante il Fondo per l'occupazione. Non possiamo inoltre non criticare la politica di taglio indiscriminato delle risorse per quanto concerne vari capitoli di bilancio, tra i quali quelli relativi al Fondo per il volontariato e contributi alle associazioni sociali (capitolo 5242), al Fondo per l'associazionismo sociale (capitolo 5246), al Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati (capitolo 3694) e soprattutto al Fondo per le non autosufficienze (capitolo 3538). Quest'ultimo capitolo viene addirittura azzerato in maniera del tutto ingiustificata e incomprensibile soprattutto in un momento di crisi in cui la garanzia dei livelli minimi di assistenza per le fasce deboli dovrebbe prioritariamente essere garantita. Con riferimento al disegno di legge finanziaria per il 2010, ribadiamo il giudizio negativo già espresso in occasione del dibattito sul DPEF: è evidente come questa manovra finanziaria 2010 leghi i provvedimenti in essa contenuti prevalentemente a risorse incerte, configurando un'impostazione sostanzialmente vincolata ai risultati di un provvedimento *una tantum* qual è lo scudo fiscale. Non possiamo qui non ricordare peraltro che i precedenti circa la validità dello strumento dello scudo fiscale al fine di drenare risorse sono assolutamente negativi. A risorse a dir poco incerte è legato anzitutto il rinnovo del contratto dei lavoratori del pubblico impiego. Di fatto, a favore dell'intero settore statale, nel triennio contrattuale 2010-2012

previsti dalla finanziaria 2010, i dipendenti statali avrebbero diritto ad un aumento di 9 euro lordi, una cifra davvero esigua che nemmeno è sufficiente al pagamento dell'indennità di vacanza contrattuale.

alla riduzione della pressione fiscale a partire dal mondo del lavoro attraverso un aumento della detrazione IRPEF per lavoro dipendente, una riduzione del prelievo fiscale sulla quota di salario e la detassazione delle tredicesime. Solo così si potrà cominciare ad uscire da questo immobilismo

per rispondere al piccolo mistero che, però, non è piccola questione: è un piccolo mistero di fronte a quelli grandi, ma non è piccola questione. Gradirei quindi una risposta su questo punto: che ne è di quei 70 milioni di euro?

378 milioni di euro stanziati nel 2009 contro i 567 previsti, ai 400 milioni di euro nel 2010 contro i 563 milioni di euro previsti

Vorrei dire che rispetto ai grandi temi della crisi economica e del suo superamento, mentre in altri Paesi cultura, innovazione, ricerca, scuola, formazione, spettacolo e beni culturali sono un volano

Signor Presidente, signor Vice Ministro, colleghe senatrici e colleghi senatori che con me condividete questo importante dibattito, penso che non dobbiamo commettere l'errore di trattare

sostanzialmente, anche negli aspetti più critici che doverosamente l'opposizione ha avanzato in questi mesi che precedono la finanziaria,

sostanziale inattaccabilità delle scelte adottate dal Governo fino a questo punto. Pur tuttavia, è importante vedere come di fronte a questa legge finanziaria si sia sviluppato un dibattito che ha coinvolto anche e soprattutto quanti tra noi avevano e hanno plaudito a queste scelte di vigore. un dibattito - beninteso - nel quale ci sono stati interventi autorevoli, soprattutto fuori da quest'Aula, in favore del prolungamento di questa politica esclusivamente di rigore: di rigore: una politica di rigore che considera non rigore qualsiasi azione di taglio ulteriore della spesa corrente o di intervento sui fondi perduti. Penso ad un autorevole commentatore come Giavazzi e ad altri interventi che si sono registrati. Eppure, nella nostra Commissione, in Parlamento, nella Commissione bilancio del Senato della Repubblica e in quest'Aula, si è sviluppato un altro dibattito, a mio avviso, importante, proficuo e con contributi che non esito a definire

all'intervento sulla cedolare al 20 per cento. Penso ad una strumentazione molto ampia che non sto qui a riepilogare perché è stata illustrata sui giornali e se ne è parlato anche negli interventi che mi hanno preceduto.

perché per ognuno di questi provvedimenti sia la maggioranza che l'opposizione hanno attentamente considerato la possibilità di gestire gradualmente una serie di iniziative che diano comunque una scossa e trasmettano l'idea che una reazione è cominciata. Sarebbe possibile portare all'interno di questo scenario di rigore rigorose reazioni, perché per ognuna di queste voci

credo con grande maturità, una possibile linea politica ed economica da intraprendere ed avviare subito, già nelle prossime settimane, dando quel segnale che il Paese si attende, si aspetta.

caso della costituzione di questo fondo sul quale far convergere tutte le economie alimentandolo con un'imposta pari al 3 per mille sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito, creando sostanzialmente una provvista fissa attraverso quest'imposta e poi una parte più variabile che dovrebbe dipendere dall'economia. Penso che nell'attesa di riuscire a stabilire un dialogo con l'opposizione su altri temi di grandissimo rilievo, quali la riforma istituzionale o quella della giustizia

di un lavoro che la maggioranza e l'opposizione hanno svolto, credo anche con grande professionalità nelle settimane che ci siamo lasciati alle spalle.

i conti pubblici registreranno un sensibile peggioramento. I capitali di investimento privati, come al solito e nonostante lo scudo fiscale introdotto, preferiranno Paesi che garantiscono maggiori certezze in termini di profitto. Nel frattempo, la rendita continuerà ad assottigliarsi e la politica industriale del nostro Paese, già evanescente, si dissolverà definitivamente. Non sono scenari pessimistici o caricaturali. Sono semplicemente proiezioni, traiettorie che la politica di questo Governo, con la complicità della maggioranza politica parlamentare che lo sostiene in ogni cosa, determineranno nei prossimi anni se non vi saranno brusche inversioni di rotta. L'immagine è quella di un Governo che, di fronte ad una crisi di proporzioni inedite, per la quale si sono sprecati similitudini e raffronti con quella drammatica del 1929, si è seduto di fronte al baratro, a contemplare la propria fragilità. Sì, l'immagine è proprio quella di un Governo fragile, a dispetto della rappresentazione mediatica che tocca sopportare e della conseguente ricaduta in termini di temporaneo consenso. La realtà, come ben sapete anche voi, è un'altra: questo è un Governo debole con i forti e odiosamente forte con i deboli; un Governo probabilmente chiamato a far fronte ad un problema più grande di sé e che si ostina a sperare che la crisi passi il più presto possibile e che tutto possa tornare come prima. È un Governo che di fronte ad evidenti scenari di particolare criticità, specie - com'è stato ricordato - sotto il fronte occupazionale, non ha saputo e voluto fare di meglio che scippare risorse alle Regioni destinate alla formazione, e non per farne l'occasione per riformare l'istituto degli ammortizzatori sociali e con essi l'intero sistema del mercato del lavoro; si è invece limitato ad estendere la cassa integrazione in deroga per tutte quelle situazioni - purtroppo tantissime e, in prospettiva, sempre di più - in cui la cassa integrazione straordinaria non era prevista. questa è una coperta che, per quanto improvvisamente allungata e spacciata per coesione sociale, è destinata a rimanere corta e leggera, inadatta a coprire e proteggere. un Governo - questo sì - molto abile e, per usare un eufemismo, pure facilitato nella sua comunicazione, che pensa di sopravvivere con una politica di annunci e spot, efficaci più per rimuovere o ottenebrare la realtà che per dare la reale percezione delle cose.

tant'è che sembra non si ponga neppure il problema. Questa quindi è una manovra che non solo non dà risposte, ma che non si pone neppure le domande necessarie. In ogni comparto dei trasporti e della logistica, manca letteralmente una visione organica animata da una logica di sistema. Governo al massimo si è esercitato, e talvolta male, nella cessione dei servizi di trasporto eserciti in regime di monopolio dal pubblico, con perdite che negli anni si sono aggravate per la mancanza di un rilancio della politica industriale di settore o per la mancanza di investimenti strategici necessari ad adeguare i servizi ai mutamenti intervenuti negli ultimi anni o più spesso per la mancata copertura dei servizi universali. La cifra che in tutta la manovra latita ed è assente è la tensione necessaria verso l'innovazione e l'ammodernamento infrastrutturale, cosa che negli altri Paesi è avvenuta e che nel nostro ha scontato significativi fattori di contrasto, da un debito pubblico che tuttora costituisce il nostro piombo sulle ali alla dispersione in mille rivoli delle poche risorse disponibili con un'atavica e anacronistica lotta di campanili, dalla vischiosità del sistema degli appalti e delle concessioni fino ai sistemi di *governance*, del tutto inadeguati a governare procedure complesse come quelle della pianificazione territoriale o della sicurezza e soprattutto rispetto alla velocità e al rigore necessari e richiesti. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: anche laddove le opere si stanno completando, con il concorso e il riconoscimento di tutti - e penso in primo luogo alla TAV, praticamente la sola opera infrastrutturale di ammodernamento del Paese negli ultimi trent'anni avviene con la triplicazione dei costi, il raddoppio dei tempi di realizzazione e il dimezzamento delle funzionalità previste originariamente. Il resto è la politica degli annunci e delle prime pietre, già vista e subita: vale per il Ponte sullo Stretto, per il MOSE o ancora per la Tirrenica e la Salerno-Reggio Calabria, solo per citare le più note. Si annuncia il finanziamento e l'integrale copertura delle opere, ma contestualmente si dilapidano risorse in progetti e piani finanziari che, nella migliore delle ipotesi, saranno buoni appunto per la posa della prima pietra, del primo pilone o del primo tratto di autostrada; dopodiché, pronti e via per l'imminente campagna elettorale del momento. Ma quanto può durare una politica così? L'Italia invece è un Paese che frana: le immagini di Giampilieri e di Messina ci hanno offerto non solo la metafora, ma direi quasi la rappresentazione plastica della situazione del Paese. Frane sistematiche si sono registrate mesi prima e sono diffuse, anche per rimanere al tema, lungo il tragitto della Salerno-Reggio Calabria che vi ostinate a dare per interamente finanziata e conclusa entro il 2012, ben sapendo di mentire scientemente a voi stessi. La realtà invece è quella di un'infrastruttura tanto necessaria al Paese quanto lasciata a se stessa, in mano - di fatto - alla criminalità organizzata, che - come abbiamo ripetutamente audito nelle Commissioni - è l'unica forza che presidia e controlla il territorio e organizza la forza lavoro. Per Giampilieri il Presidente del Consiglio si è affannato a declamare il modello Abruzzo, dove gli *spot* televisivi di tanto in tanto fanno vedere sistematicamente la consegna di qualche casetta di legno, senza mai dare voce e visibilità alle condizioni di vita grame della stragrande maggioranza della popolazione, che vive ancora nelle tende. È l'ora invece, a parer mio, di accendere i riflettori anche su di loro. Nell'attesa di comprendere quale sia effettivamente il modello Abruzzo che viene inteso, registriamo che per la tragedia ferroviaria di Viareggio, al di là dei proclami e delle circostanze di rito, niente si è fatto per i congiunti e i familiari delle vittime, né per il ripristino delle condizioni abitative distrutte. Visto che nella manovra finanziaria non c'è un euro "sonante e ballante" sarebbe opportuno che ci segnalaste le vostre reali intenzioni su un'ipotesi di apposita legge speciale, ventilata nei mesi scorsi ma di cui, a parte la nostra iniziativa parlamentare, non si scorge traccia. Noi intanto abbiamo presentato anche un ordine del giorno al riguardo e preghiamo i colleghi della maggioranza di condividerlo, disponibili ovviamente a rivederne le forme e i toni. Dal punto di vista delle infrastrutture, la situazione sta diventando ormai grottesca. Non solo non si aggiungono risorse e non si liberano quelle già stanziate, ma addirittura si assiste ad una situazione in cui il Ministro dell'economia mette le mani in tasca al Ministro delle infrastrutture e questi cerca di rifarsi sugli utenti dei servizi, ritoccando sensibilmente le tariffe, senza in cambio neppure la garanzia di migliorare i servizi stessi. Fuor di metafora, nella finanziaria alcuni capitoli non banali per la realizzazione di infrastrutture ferroviarie e stradali, nella disponibilità del Ministro dell'economia, sono stati dimezzati o letteralmente azzerati per un importo complessivo superiore ai 3 miliardi di euro.

Signor Presidente, la vera novità di questa finanziaria snella è per l'appunto, come diceva prima il collega Augello, il dibattito che è si è aperto sul resto, cioè su quello che bisognerebbe fare per affrontare la crisi e soprattutto (questa è la novità di fondo) su come coprire queste ricette, cioè su come tagliare la spesa pubblica. È la prima volta, forse, in cinquant'anni che vediamo gli uffici lavorare sulle possibilità e sulle modalità di taglio della spesa pubblica e non sull'invenzione di modi per spremere i contribuenti (quindi per aumentare le tasse), per poi fare qualcos'altro. Come si è arrivati a questa situazione lo sappiamo tutti. Adesso le ricette sono varie, diverse e modulabili; non ripeto gli argomenti già detti, dall'IRAP alla cedolare sugli affitti, ad un intervento a favore delle famiglie. Tutto questo si vedrà nel corso dell'*iter* della finanziaria. Il punto chiave è che forse - sottolineo forse - è arrivata anche nel Palazzo la consapevolezza che bisogna cambiare registro. Due conti semplici: uscite 800 miliardi, entrate 720 miliardi. Peccato che la macchina pubblica stia in piedi con le entrate del settore privato; quindi la macchina pubblica non potrà andare avanti in eterno ad avere 800 miliardi di uscite se non ci sono le entrate per coprirle. Questo è il dato di fondo. Anche perché noi abbiamo avuto un tracollo delle entrate. Il buco previsto era di 30 miliardi circa e adesso è di 80 miliardi; nell'anno venturo si prevede più o meno di rimanere nella stessa condizione. Ma siamo sicuri che l'anno venturo entreranno 720 miliardi di euro?

Quindi ci scontreremo con una spesa pubblica che va come su un binario parallelo, in una realtà distinta dal mondo reale, e con entrate che invece

E allora cosa fa l'azienda Italia? Questo secondo noi è il dato interessante. Se una normale azienda privata ha un calo di fatturato, tira la cinghia, razionalizza la spesa, i premi del personale si riducono all'osso

La cassa integrazione non esiste per definizione; figuriamoci parlare di mobilità e licenziamento per enti in sovrannumero! Il punto è: fino a quando si riuscirà a sostenere questa situazione? Per questo motivo insistiamo su riforme

Allora, ragioniamo su qualità e quantità di spesa e dei servizi erogati; anticipiamo finalmente il ragionamento sui costi standard. standard. Farò tre esempi banali: servizi pubblici locali, giustizia e scuola; si tratta di tre fattori fondamentali per la competitività del sistema Paese.

nemmeno fare un'ipotesi di razionalizzazione; essa non può matematicamente stare in piedi. È evidente che si tratta di realtà dove ci sono fortissimi margini di miglioramento, di taglio e di razionalizzazione della spesa. Quanto il *World economic forum* ha evidenziato come il principale fattore di non competitività del sistema Italia sia costituito non tanto dalle tasse, come si pensa; paradossalmente, per le imprese è peggiore l'inefficienza e il peso della burocrazia. La giustizia è un esempio eclatante: su 134 Nazioni, l'efficienza del sistema giustizia Italia è al 124° posto. Ci superano forse il Paraguay, l'Uruguay e qualche Stato del Centro Africa. Allora si dirà: spenderemo poco per la giustizia. Non

si spende di più e si è al 124° posto, qualcosa non quadra. È evidente che la giustizia è un altro settore dove ci sono ampi e fondamentali margini di razionalizzazione, di taglio e di miglioramento della spesa.

per risolvere il problema scuola si dovesse assumere più personale. Ma non è questo il punto: non dobbiamo assumere più personale, ma avere personale preparato. Andiamo dunque a verificare se la nostra scuola funziona.

che maturano nel mondo, probabilmente troveremo anche il modo di far lavorare le persone. Ogni tanto, poi, la maggioranza e il premier richiamano il «miracolo di Napoli»

presentando gli emendamenti. Mi auguro che su quello che abbiamo evidenziato, su queste poche parole che ho detto e su quello che abbiamo scritto nell'intervento e su cui insieme abbiamo cercato di lavorare

Signor Presidente, signor Vice ministro, onorevoli colleghi, questa finanziaria è attenta ad assecondare lo sviluppo, senza far crescere il debito pubblico. La scelta fatta da Tremonti di rigore nei conti pubblici non può che essere condivisa. È in gioco la credibilità stessa del Sistema Italia. Al di là di questo, tuttavia, credo che vada fatto un ragionamento politico più ampio. Voglio subito complimentarmi con la Commissione bilancio per il dibattito serio ed approfondito che lì si è svolto e con il relatore

credo che con una maggioranza così ampia e leale come quella che sostiene il Governo, noi si debba saper anche rappresentare uno stimolo nei confronti del Governo stesso, come si fa d'altro canto in tutte le democrazie mature;

i timori di mettere sul tavolo ulteriori problematiche, di offrire ulteriori soluzioni a questo Governo. Governo. Al di là di quanto fatto, che non può che essere condivisibile, ritengo che sia questo il momento in cui dobbiamo accelerare la ripresa, iniziando a realizzare proprio ora il nostro programma elettorale. In particolare, dobbiamo avviare il taglio delle tasse sulle imprese e sulle famiglie, tema che ha costituito uno dei fondamenti della nostra campagna elettorale

Dobbiamo trovare le risorse, ovviamente non aumentando l'indebitamento ma sottraendole alla spesa improduttiva; dobbiamo trovare delle risorse

il ministro Tremonti quando ha inserito tra le priorità dello scudo fiscale la ricerca e l'università. Si parla di una restituzione di risorse per circa 400 milioni di euro. va detto anche con grande onestà, di un intervento *una tantum*. Occorre invece, a mio avviso, una strategia che tenga conto, peraltro ovviamente, della criticità del momento. Tutti i principali Paesi, dagli Stati Uniti, alla Francia, alla Germania, proprio in questa congiuntura hanno deciso

eccellenza. Da qui alcune proposte che con alcuni colleghi abbiamo avanzato in questa finanziaria; innanzi tutto il finanziamento di 10 strutture di eccellenza, come si è fatto in Germania e come si sta facendo in Francia, proprio per dare al nostro sistema universitario, quello che è probabilmente ancora oggi l'*handicap* maggiore, centri che possano essere fortemente competitivi a livello internazionale. Investire dunque sulla qualità. Collegare poi ancora l'impresa all'università. di deduzione fiscale coloro che investono in società finalizzate al finanziamento di progetti di ricerca *high-tech,* ed ancora, l'individuazione di risorse che possono derivare da contribuzioni aggiuntive

per favorire i prepensionamenti degli insegnanti anziani in modo da consentire l'assunzione degli insegnanti precari. Questo emendamento è stato dichiarato inammissibile; conto di riproporlo in altra sede.

c'è necessità di dare invece spazio ed energie fresche e nuove. Oltretutto un'iniziativa di questo tipo non avrebbe un costo significativo per l'erario e consentirebbe di risolvere un gravissimo problema sociale come quello del precariato della scuola.

che non sempre si può risparmiare; chi vuol sempre risparmiare è perduto». Si tratta di una massima esemplare, che tuttavia va resa compatibile con le risorse di cui si dispone, o che si ritiene di poter recuperare sulla base di specifici provvedimenti. Ebbene, credo che la legge finanziaria ed il bilancio che stiamo discutendo tengano bene in conto sia la massima di Fontane, sia il suo presupposto cui facevo riferimento. Si tratta di un testo snello che non tralascia di affrontare alcune questioni speciali che da tempo vengono discusse in questo Parlamento e che affronta anche questioni di minore entità e che tuttavia costituisce un modello di transizione in vista della riforma della legge di contabilità

lavoro svolto dal Governo e dalla Commissione desidero soffermarmi su alcune questioni contenute negli emendamenti firmati dal sottoscritto e da altri colleghi, che si rivolgono ad una riduzione del carico fiscale, alla formazione di maggiori entrate e di minori spese, così da attrarre, mi auguro, l'attenzione del Governo su temi che appaiono maturi per essere trattati dal Parlamento stesso. Mi riferisco al taglio dell'IRAP, cui è necessario pensare al di là degli schieramenti interni ed esterni alla maggioranza; mi riferisco all'opportunità di prorogare i termini di definizione dello scudo fiscale per le operazioni scaturenti da vendite immobiliari o azionarie; mi riferisco all'annosa e paradossale questione delle case da gioco; mi riferisco, infine, alla necessità di ampliare l'effetto della cosiddetta «rottamazione del pubblico impiego» cui anche il collega Valditara, relativamente alla scuola, faceva riferimento, ed alla piena attuazione delle previsioni della legge n. 133 del 2008 in materia di cessione delle partecipate. Con il taglio dell'IRAP si offrirebbe una boccata di ossigeno al sistema imprenditoriale e dunque al drammatico tema dell'occupazione, particolarmente avvertito nel Mezzogiorno. Con la proroga dei termini per lo scudo fiscale per le operazioni accennate si aumenterebbe, e non di poco, il rientro di capitali e delle relative tasse a ciò connesse. Altro che tutele di chissà quali loschi affari: qui ci sono 300 miliardi di euro italiani all'estero. Se vogliamo farne a meno possiamo anche discuterne, ma sicuramente non sarebbe nell'interesse del Paese. Con la vicenda dei casinò, cui facevo riferimento prima, si rilancerebbe il turismo in zone di crisi e si accrescerebbero le entrate dello Stato. Con la rottamazione del pubblico impiego, come è prevista dall'articolo 72 della legge n. 133 del 2008 che verrebbe prorogato di un anno, si risparmierebbero notevoli risorse e si alleggerirebbe l'apparato burocratico, come attesta la relazione tecnica della Ragioneria. Con la cessione delle quote delle partecipate si farebbe cassa e si attenuerebbe il triste fenomeno della gestione clientelare delle stesse. Vi è un ultimo elemento che vorrei porre all'attenzione del Governo relativamente alla gestione dei singoli rami dell'amministrazione dove ancora, nonostante gli interventi dei vari Ministeri e del ministro Brunetta in particolare, si registrano duplicazioni ed autoreferenzialità del tutto tutto incompatibili con le condizioni dei conti pubblici e con il principio del federalismo fiscale. Il presidente Berlusconi dice spesso che difficilmente i tacchini sono disponibili ad anticipare il Natale: è vero, ma nei Ministeri, nelle Regioni, negli enti locali e negli enti pubblici in genere ci sono ancora

ed accelerare la ripresa, il Mezzogiorno ha bisogno di lavoro e di infrastrutture, l'amministrazione pubblica di efficienza, trasparenza e responsabilità. La finanziaria che stiamo discutendo offre solo alcune risposte, quelle più urgenti, e questo è importante; ma bisogna fare di più, molto di più, con coraggio e determinazione perché, come diceva Guicciardini, non basta la prudenza nelle spese, è necessario saper spendere con vantaggio e nell'interesse del Paese che è fatto di Nord, di Centro e di Sud, di emergenza e di povertà, non certo di teatrini e spaccature politiche su scelte